è prima di tutto l'occasione per rendere un ulteriore omaggio, da parte dell'Assemblea del Senato,

a Maria Riboli, a Cristian Rossi e a Marco Tondat.

Nove nostri concittadini, nove vittime del terrorismo, che l'Italia non dimenticherà. Venerdì scorso, alle 21,10, la nostra ambasciata veniva informata dell'attacco in corso all'Holey Artisan Bakery. A chiamare era Gian Galeazzo Boschetti, marito di Claudia D'Antona. Boschetti informava che, dopo essersi allontanato momentaneamente dal tavolo verso il giardino, aveva visto irrompere, attraverso il giardino, quattro o cinque individui armati. Verso le 21,45, quindi una mezz'ora dopo, si metteva in contatto con l'ambasciata un altro connazionale, Jacopo Bioni, *chef* di cucina, che attraverso la scala del retro della cucina aveva raggiunto il tetto e da lì il giardino, allontanandosi e trovando rifugio presso un'abitazione privata. Nel frattempo, il primo intervento della polizia si era concluso con un insuccesso, con l'uccisione di due ufficiali e il ferimento di una ventina di altri poliziotti per l'effetto di lancio di granate. Successivamente, Boschetti comunicava che dalla posizione in cui si trovava, nascosto in giardino, vedeva due o tre membri del commando terroristico sorvegliare l'area, sia dal terrazzo del secondo piano che dalla sala del piano terreno, dove erano stati raccolti la maggior parte degli ostaggi, e sentiva ad intervalli irregolari raffiche di mitra. La mattina dopo, alle 7,42 di sabato 2 luglio, è scattata l'operazione condotta dall'esercito, con il dispiegamento di quindici mezzi corazzati, due dei quali hanno sfondato la rete di recinzione e la parete d'ingresso del locale. L'intervento è durato una decina di minuti per lo sfondamento, mentre l'operazione nel suo insieme, che ha comportato naturalmente anche la bonifica (con il brillamento degli esplosivi) del teatro dell'attacco terroristico e della presa degli ostaggi, è durata circa quaranta minuti. Il riconoscimento delle vittime (delle nove vittime italiane, delle sette vittime giapponesi e degli altri) è avvenuto lo stesso sabato 2 luglio, alle 18 ore locali, nell'obitorio militare. Il riconoscimento confermava subito che alcune vittime erano decedute per colpi di arma da fuoco, mentre per le altre il decesso era dovuto a colpi di macete inferti al collo, alla nuca e al volto. Una lunga notte di orrore e di agonia dunque, nel corso della quale l'ambasciata è stata continuamente in contatto con l'unità di crisi e quest'ultima con le famiglie, la cui presenza nel ristorante era stata nel frattempo accertata e che, naturalmente, continuavano a sperare. Gli autori di questo infame massacro erano giovani istruiti, appartenevano a famiglie della classe media e alcuni addirittura dell'*establishment* bangladescio, così smentendo - e non è la prima volta - facili interpretazioni sociologiche del fenomeno terroristico contemporaneo al quale siamo di fronte. Secondo le autorità locali, si tratterebbe di aderenti al gruppo islamico Jamaat-ul Mujahideen. Le nostre prime valutazioni, che abbiamo fatto anche con colleghi diplomatici e dell'*intelligence* di altri Paesi, portano comunque a ritenere attendibili le rivendicazioni della strage fatte da Daesh in alcuni siti del sedicente Califfato. Onorevoli senatori, questa tragedia credo che proponga alla nostra attenzione e al nostro dibattito alcune valutazioni. Anzitutto sul carattere della minaccia, sul fatto che siamo di fronte ad una minaccia globale, che dall'Africa occidentale si spinge fino al Sud-Est asiatico, dal Golfo di Guinea al Golfo del Bengala, che ha forme diverse, Daesh, Al-Qaeda, diversi gruppi jihadisti locali, ma che ha un comune denominatore nella degenerazione del fondamentalismo terrorista di di matrice islamista e che ha in comune anche la capacità simbolica di attrazione di Daesh.

certo in questo caso le vittime sono state prevalentemente, anche se non esclusivamente, italiani e giapponesi. In altri casi i bersagli sono stati comunque bersagli identificati come infedeli; occidentali, stranieri, quelli che il terrorismo folle e omicida definisce infedeli. E spesso i bersagli - dobbiamo dircelo con altrettanta chiarezza - sono nel mucchio; si spara nel mucchio. La strage più cruenta è stata quella di tre giorni fa a Baghdad, con la morte di oltre 200 persone. Si spara quindi nel mucchio e si spara nel mucchio anche in Paesi a maggioranza musulmana. Quindi, certo che noi siamo bersagli, lo siamo in quanto italiani, lo siamo in quanto occidentali, lo siamo in quanto difensori dei valori delle nostre società. però altrettanto certo che il terrorismo colpisce spesso anche in modo indiscriminato e prende a bersaglio anche Paesi a maggioranza islamica.

che deve essere, io credo, innanzitutto una risposta di unità del Governo, del Parlamento, delle istituzioni coinvolte, delle forze sociali e del mondo della cultura. Quando uccidono nove connazionali, l'Italia risponde unita. E questo deve essere, credo, un messaggio che diamo in modo molto chiaro.

che il terrorismo fondamentalista, a maggior ragione dopo questa strage, non avrà tregua da parte nostra. Dacca ci dice che la risposta alla minaccia terroristica è necessaria e deve essere decisa. Si dice che con questi attentati Daesh risponda con il terrorismo alle sconfitte che sta subendo sul terreno. Io dico una cosa molto semplice, e cioè che solo la mobilitazione internazionale per la sconfitta definitiva di Daesh può cancellare l'attrazione simbolica che oggi è il motore principale che attiva questi attentati. Dobbiamo essere convinti di questo, perché se interiorizzassimo quasi un discorso di incertezza o di paura nel proseguire e condurre fino in fondo il contrasto a Daesh, immaginando che una certa riluttanza nel contrasto a Daesh potrebbe risparmiare qua e là, in giro per il mondo, o nei nostri confini nazionali, ci sbaglieremmo di grosso, perché è l'esistenza di Daesh che produce l'attrazione simbolica che è alla base di queste azioni infami. Cellule organizzate o lupi solitari, gruppi locali o cani sciolti: non sappiamo bene questo gruppo dei cinque che ha attaccato il ristorante di Dacca di quale di queste categorie faccia parte. Ma tutti spesso compiono i loro gesti criminali in nome del richiamo a questo sedicente Stato islamico. Quindi abbattere questo simbolo resta un obiettivo fondamentale del Governo, del Parlamento e dell'Italia. Naturalmente non basta vincere sul piano militare e l'Italia lo va ripetendo, come sapete, da mesi nell'ambito della nostra coalizione internazionale e con i nostri alleati. Non basta perché sappiamo che il contrasto alla radicalizzazione fondamentalista sarà comunque un impegno di lunga durata. Sconfiggere Daesh sarà un passo decisivo, ma non definitivo, ed è qui credo che dobbiamo offrire solidarietà e chiedere impegno ai Governi dei Paesi a maggioranza islamica e alla comunità islamica in Italia. Offrire solidarietà, perché molto spesso sono loro gli obiettivi e i bersagli del terrorismo, e Baghdad, per citare solo l'ultima strage, ce lo ricorda. Ma anche chiedere impegno, perché, come ripete spesso uno dei *leader* del mondo arabo, re Abd Allah di Giordania: «Tocca a noi, a noi arabi, a noi credenti nella fede islamica battere questi infedeli». Così li definisce re Abd Allah. Ed io mi rivolgo da quest'Aula e con questo spirito di solidarietà e di richiesta di impegno anche alla grande, vasta comunità musulmana che vive in pace nella stragrande maggioranza del nostro Paese, chiedendo anche a voi, anche in Italia, di impegnarvi a viso aperto, unitariamente, contro questi terroristi che abusano della vostra religione deturpandola. La vostra mobilitazione e il vostro impegno saranno decisivi nell'attività di contrasto alla radicalizzazione, di isolamento e di sconfitta del terrorismo.

di Cesare Tavella, un altro italiano, un cooperante ucciso anche lui in Bangladesh lo scorso mese di settembre. I nostri nove connazionali non erano in vacanza (non c'è niente di male ad essere in vacanza, naturalmente) e non erano in un nuovo Eldorado. Avevano scelto di lavorare in Bangladesh, un Paese, specie nel settore tessile, nel quale lavoravano queste nove persone, ricco di potenzialità, ma anche di enormi contraddizioni. Paese in cui, nel tessile in modo evidente, potenzialità di sviluppo e contraddizioni della povertà si intrecciavano e si intrecciano in modo drammatico. drammatico. Basti ricordare, come molti hanno ricordato in questi gironi, il crollo del Rana Plaza nel 2013. crollo di un edificio sotto le cui macerie furono trovate 1129 persone. Quasi tutti, molti di loro, lavoravano in condizioni certamente non di sicurezza in fabbriche tessili di vario genere. essi avevano scelto un Paese e un settore nel quale era evidente l'intreccio tra grandi potenzialità, ma anche grandi difficoltà e contraddizioni sociali. E avevano fatto questa scelta in un Paese in cui da anni erano evidenti, evidenti, segnalati dalle diverse cancellerie e diplomazie internazionali, rischi crescenti di instabilità. C'erano stati dei segnali premonitori, che continuano ad esserci. Avrete visto che questa mattina c'è stato di nuovo un attentato, in occasione della fine del Ramadan, proprio in Bangladesh. Lì avevano scelto di andare a lavorare. Alcuni lo avevano fatto per spirito d'impresa, anche successo nel loro lavoro come imprenditori. Altri, semplicemente, lo avevano fatto per cercare quel lavoro che non avevano trovato nel nostro Paese. E ce lo siamo sentiti dire dai loro familiari Persone diverse, ma accomunate, tuttavia, da spirito di iniziativa, da creatività, da capacità di stare con gli altri, da generosità, da attaccamento alla famiglia e ai nostri valori. Abbiamo perso nove persone dotate di queste qualità. Nove italiani.

abbia inizialmente definito la sua informativa come una ulteriore occasione perché il Senato possa rendere omaggio alla memoria di questi nostri nove concittadini. L'attacco è stato particolarmente vile e, nella ricostruzione che il Ministro ha dato, particolarmente drammatico, considerando quel Boschetti che dal giardino era già in contatto la nostra ambasciata. L'attacco, però, ci deve portare a fare alcune considerazioni, non soltanto cronistiche. La prima, signor Ministro, che lei ha giustamente sottolineato, il reclutamento di questi terroristi. Mi pare che da lei siano state citate con diffidenza, se non con insofferenza, tante stupidaggini sociologiche

dai ceti dirigenti, in taluni casi dallo stesso *establishment* di certo mondo. La rivendicazione, più che credibile, è pervenuta dall'odioso Daesh. Certamente la guerra contro questi avversari deve avere un carattere internazionale e globale, come giustamente lei ha detto a proposito della minaccia. Ma dobbiamo stare attenti, perché è vero che nella sconfitta sul terreno di guerra, guerriglia e terrorismo c'è una certa continuità e contiguità fra i tre territori di sfida. Sarà un momento decisivo, ma non per questo un momento definitivo, nel senso che vincere questa guerra implica, la solidarietà e l'impegno delle vaste comunità islamiche che in Occidente vivono in pace. Sì, ma è troppo generale e troppo generico questo suo riferimento. A noi sembra invece, fin dalle parole del Presidente egiziano all'indomani del drammatico episodio di Parigi, l'assassinio di Charlie Hebdo, che bisogna chiedere l'impegno di queste strane figure a cavallo tra l'universalismo della fede e l'esasperazione fondamentalista e nazionalistica. Il Presidente dell'Egitto in quelle vacanze di Natale che precedettero di una decina di giorni

abbiamo tutto il mondo in guerra con noi". Fu un discorso importante, importantissimo. A vergogna della stampa occidentale questo discorso è entrato in circolazione nelle nostre considerazioni soltanto dopo

a tutta la vastissima comunità islamica, che vuole vivere in pace e che è minacciata non meno di noi

Ho l'impressione che dobbiamo ripensare molti nostri comportamenti anche istituzionali proprio alla luce delle sue considerazioni, Se lei vuole servirsi della giornata di oggi per chiedere al Senato e all'arco parlamentare la massima unità di intenti e di azione, con un Gruppo come il nostro, collocato all'opposizione, ma mai all'opposizione della politica internazionale del proprio Paese, lei sfonda una porta aperta. però accentuare certi collegamenti internazionali che abbiamo trascurato. Signor Ministro, quando il terrorismo fondamentalistico - parlo di qualche decennio fa - aveva un unico bersaglio, lo Stato di Israele, quel terrorismo era egualmente odioso, ma il nostro Paese pensò, con autentica miopia nei rapporti internazionali, di poter coabitare, negoziare e neutralizzare con esso in qualche modo. Oggi questo terrorismo lei l'ha chiamato islamico; io mi permetterei di darle un suggerimento che viene dalla storia di questa Assemblea: il senatore Benedetto Croce, dopo il delitto Matteotti, non usò più l'aggettivo «fascista», ma «fascistico». Per quel che vale, questo è un fondamentalismo «islamistico», che deve portarci ad accentuare la nostra avversione e la nostra avversità, anche sul terreno. Ho avuto l'onore di accompagnare il presidente della Commissione affari esteri, il senatore Casini, in una missione sul terreno nel Kurdistan iracheno. La sensazione è che lì le cose stiano volgendo a vantaggio a vantaggio della coalizione della quale ci onoriamo di far parte. Ma, proprio per questo, è da mettere nel conto - e purtroppo è arrivata - una recrudescenza sempre più odiosa di questo terrorismo islamistico che, come lei ha detto, si rivolge contro gli infedeli. Da questo punto di vista, non manchiamo di lealtà alla memoria dei nostri concittadini se anche noi, di fronte a tutto questo, non possiamo non sentirci infedeli, a prescindere dalla nazionalità dei caduti. *(Applausi dai

di trovarci a discutere in maniera approfondita di questi temi. Credo che sia necessario chiamarlo terrorismo islamista o islamico, comunque, perché è un dato di consapevolezza; lo è per noi tutti, per la comunità occidentale, ma lo deve essere, in senso di stimolo, anche per le comunità che sui nostri territori si riferiscono a quella religione. La consapevolezza diventa realtà e la realtà diventa reazione e la loro reazione diventa essenziale per arginare, almeno sui nostri territori, con la loro collaborazione (che fino ad ora forse non è stata complessiva e completa),

nel momento in cui ha capito che stava cadendo il sogno accarezzato per un paio d'anni di un neo-ottomanesimo, tanto che alcune azioni sono state palesi: la Turchia cercava infatti di indirizzare la sua area di influenza sia verso la penisola balcanica storica, sia verso i Paesi che guardano verso Sud.

Paese ci ha fatto rischiare un'*escalation* quando ha abbattuto un aereo russo. Non entro nei particolari, ma penso che lei abbia vissuto come noi la preoccupazione del richiamo che la Russia e la Turchia si trovassero in una situazione di belligeranza

anche concreto: abbiamo visto con quanti attori si svolge quella situazione difficile e non dobbiamo dimenticarne nessuno. Noi abbiamo sicuramente

quegli stipendi e quei funzionari hanno bisogno di finanziamenti e per quello le dicevo che nel loro autoriconoscimento come Stato c'è un passaggio ulteriore. Notizie conosciute riferiscono che in pochi anni dai Paesi sauditi, anche attraverso fondi sovrani,

considerazioni che forse possono sembrare dure, ma penso che si inseriscano nella risposta ferma della comunità occidentale, non solo italiana, a questa situazione.

Signor Ministro, queste cose non le sapremo mai, però andrebbero fatte. Forse è il caso di cominciare a dirle a questi signori malvagi e cattivi, che sicuramente non rappresentano nemmeno la loro stessa civiltà. Presidente, signor Ministro, avevo chiesto la sua presenza e abbiamo avuto ragione perché quella di altri rappresentanti, ancora più titolati, avrebbe rischiato di

Il nostro Paese, inserito nel contesto occidentale, ha una lunga tradizione, al di là dei comportamenti talvolta eccessivi

nel Centro Africa fu tale per cui nei decenni successivi la visione del mondo occidentale nei confronti del Centro Africa cambiò totalmente.

se non l'immediata soluzione, una comprensione che determinò una successiva fase di rapporti tra il Nord Africa e l'Europa, che non ha più registrato ulteriori simili nefandezze. Da un lato, sono portato a valutare con attenzione e gratitudine l'intervento; dall'altro - mi rivolgo in questo caso alla maggioranza - ho una grande preoccupazione, e cioè quella che il Governo non sia capace di inserirsi, nella sua apicalità, in un contesto di ragionamento del mondo occidentale, che richiami quelli che dovrebbero essere gli alleati di quel mondo ad un'azione complessiva che possa portare ad una reazione determinata e conclusiva di questa fase incredibile, nella quale si parla troppo.

valutata attraverso il «politicamente corretto»; in questo caso, si hanno reazioni come la Brexit, il successo di Trump e la considerazione scarsa che il mondo

la puntuale ricostruzione dell'eccidio da parte del ministro Gentiloni Silveri dovrebbe indurre tutti, in questa gravissima contingenza, a concentrarci esclusivamente sul rinnovato cordoglio e sulla difesa dell'interesse nazionale, nella consapevolezza ormai comune che la guerra in atto riguarda anche noi. Da parte del Governo ci aspettiamo un atteggiamento rigoroso per pretendere dalle autorità bengalesi la massima chiarezza sul perché non c'è stata una cooperazione efficiente nella gestione di questa tragica vicenda; ma questa non è una polemica, perché non è il momento delle polemiche. Il terrorismo islamico rappresenta infatti una minaccia globale e l'Italia è in prima linea così come tutto l'Occidente. Un Occidente che ha commesso errori strategici nel fronteggiare questa guerra asimmetrica che ora l'Europa chiama minaccia ibrida e sta prendendo le necessarie contromisure per la sicurezza interna ed esterna con un'agenda di contrasto che, però, prevede come sempre in questa Unione europea - tempi di reazione troppo lunghi, perché si parla di metà 2017. La minaccia, però, è terribile e attuale e va fronteggiata subito con i mezzi più idonei. L'Italia ha difeso la sua dignità nazionale dopo dopo l'assassinio di Giulio Regeni, richiamando l'ambasciatore dal Cairo e poi sospendendo le forniture per gli F-16 all'Egitto. senza rinunciare alla ricerca della verità, sarebbe un errore drammatico non porre fine a questa *escalation* negativa nei rapporti con un Paese strategico nella lotta al terrorismo. modo, va subito ripreso il progetto di collaborazione anti-terrorismo tra la NATO e la Russia, altro *partner* cruciale in questa guerra.

non lo è Daesh, non lo è Al Qaeda e non lo sono i loro seminatori di morte, quasi tutti figli dell'alta borghesia dei Paesi islamici o di famiglie già integrate da tempo in Occidente. l'equazione immigrazione uguale terrorismo è quantomeno forzata, anche se a fronte di una migrazione di queste proporzioni è lecito pretendere un controllo più severo delle nostre frontiere, che sono anche quelle europee. In secondo luogo, il terrorismo islamico colpisce indiscriminatamente non solo gli occidentali e i cristiani, ma anche i musulmani che non accettano la violenza e il terrore. È però lecito pretendere dal mondo islamico cosiddetto moderato una presa di distanze molto più forte e convinta. l'ISIS sta perdendo terreno a livello militare in Siria, Iraq e Libia. Il Califfato si decompone e questo lo induce ad adottare lo schema originario di Al Qaeda: seminare il terrore fra noi nel tentativo di creare *caos* e dividerci. chiudersi in nazionalismi esasperati che minano l'unità delle democrazie sarebbe la risposta più sbagliata. credo sia necessario riflettere sul fatto che mentre l'offensiva del terrorismo islamico è in pieno svolgimento, il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti non avrebbero dovuto destabilizzare l'Iraq e che il mondo sarebbe migliore se dittatori come Saddam Hussein o Gheddafi fossero ancora al potere. un'analisi superficiale e inesatta, perché i conflitti nel mondo islamico non sono stati creati dall'Occidente e l'ISIS non è nata per colpa nostra. Bisogna altresì riflettere sul fatto che la Gran Bretagna, con il rapporto Chilcot, sta mettendo sotto accusa l'ex *premier* Tony Blair proprio per la guerra del 2003 in Iraq e proprio mentre l'offensiva del terrorismo islamico è al suo apice. forse di un insensato segno di debolezza o, forse, è invece questa la vera forza dell'Occidente: la forza delle democrazie che possono sbagliare, ma poi sanno mettersi in discussione, a differenza dei regimi teocratici. È anche vincendo questa battaglia culturale, che deve coinvolgere il mondo musulmano, che si può avere ragione sul terrorismo islamico.

e, sotto il profilo globale, coloro che nei Paesi arabi, in Africa o in altri scenari regionali si oppongono alla strategia sanguinaria dell'ISIS. Nel contempo, l'assassinio di nove nostri connazionali e delle altre vittime a Dacca presenta aspetti in parte mai conosciuti fino ad oggi, che impongono ulteriori riflessioni. È infatti indispensabile soffermarsi sulla natura non casuale delle vittime italiane quale obiettivo primario dell'azione terroristica a Dacca, seppure (come da lei affermato, signor Ministro) occorre essere chiari in merito al fatto che «la follia terroristica vede in generale negli occidentali e negli stranieri un bersaglio». È fondamentale riflettere sul fatto che l'attentato di Dacca associa un'ulteriore modalità di attacco alle molteplici identità e tecniche che sono il tratto distintivo dell'ISIS, delle sue cellule e dei suoi adepti di ispirazione jihadista nei diversi scenari geopolitici di crisi e nelle aree regionali più esposte. In altri termini, la dinamica e gli autori dell'attentato di Dacca possono configurare, allo stato delle informazioni, una realtà ancor più complessa della sfida terroristica. uno scenario globale nel quale sono contestualmente presenti cellule parte dell'organizzazione terroristica dell'ISIS, gruppi locali addestrati dall'ISIS, che si richiamano agli obiettivi ed all'ideologia totalizzante dell'islamismo radicale e, infine, cellule e kamikaze locali e del tutto autonomi, che concorrono a diffondere e realizzare la guerra dell'ISIS o, più in generale, la follia terroristica, ma che non possono essere assimilate all'ISIS o ad altre potrebbe essere la più accreditata nell'attentato di Dacca, ma ciò che è ormai fondamentale comprendere è che alla strategia terrorista dell'ISIS è inevitabile associare natura, autori e tecniche di terrore molteplici e differenti. Anche per questa ragione condividiamo l'impegno del Governo, del Presidente del Consiglio e suo, signor Ministro degli affari esteri, sia in sede europea, sia nel confronto avviato nei diversi organi internazionali, sia nel rapporto con la Russia, in ordine alle posizioni e alle politiche che è indispensabile porre in essere al fine di superare le carenze e i ritardi della strategia occidentale nei confronti dell'ISIS. Occorrono strategie unitarie e globali in risposta al terrorismo dell'ISIS o di altre realtà che appartengono all'islamismo radicale, in primo luogo da parte dell'Unione europea, degli Stati Uniti, dei Paesi occidentali, della Russia, ma anche da parte dei Paesi o delle comunità che nel mondo arabo sono oggetto della guerra posta in essere dall'ISIS e da altre realtà che sono o si identificano nei jihadisti. Non vi possono essere risposte unilaterali che si richiamano ai diversi interessi nazionali e che, per questa ragione, i singoli Paesi ritengono più opportune. Sotto il profilo strategico è stata e sarebbe una visione parziale, frammentata, debole, priva di una visione efficace. È sostanzialmente lo scenario entro il cui l'ISIS si è sviluppato, come organismo di terrore e soggetto militare che investe i confini e i territori della Siria e dell'Iraq. Non vi sono quindi strategie esclusivamente nazionali possibili: o la risposta è dell'Europa, di un'Europa integrata, che sia soggetto di raccordo tra la NATO e la Russia (come pure è stato affermato dal Governo), o la strategia univoca, senza tentennamenti, globale, non solo militare, unitaria, o altrimenti non vi sono margini e opportunità di contrapporsi con successo alla follia terroristica.

anzi, per dirla tutta, quasi tutti. Lo dico perché spiace che un collega non abbia ritenuto di doversi alzare e rendere omaggio ai nostri connazionali uccisi. Questi atteggiamenti non vanno nella direzione dell'unitarietà della risposta nazionale alla minaccia terroristica. Però, mettendo da parte ogni polemica (sinceramente non è il momento), la ringrazio, signor Ministro, per la sua informativa, che condividiamo.

nelle occasioni passate in cui ci siamo trovati a piangere morti in molti posti del mondo, abbia saputo usare parole misurate ed abbia impostato

non dobbiamo illuderci del fatto che questa lotta per sconfiggere Daesh sia breve e rapida. Dobbiamo sapere che la guerra asimmetrica di cui stiamo parlando probabilmente continuerà anche quando, speriamo presto, la sconfitta di Daesh sarà un fatto compiuto. Naturalmente voglio anche dire con grande forza a quest'Assemblea che noi davvero siamo chiamati ad uno sforzo straordinario, ad un impegno grandissimo, politico, ma anche culturale: quello di sapere che dobbiamo sconfiggere Daesh,

Battere Daesh significa esattamente non rinunciare a quanto le democrazie dei nostri Paesi hanno costruito in questi anni.

e una possibilità di attraversare le grandi questioni del nostro tempo senza che la guerra diventasse l'unico orizzonte possibile. Signor Ministro, voglio però anche dire (ed è anche su questo che credo vada fatta una riflessione seria pacata che però metta al centro del dibattito alcune questioni di cui probabilmente abbiamo discusso poco in questi anni) che per sconfiggere Daesh dobbiamo interrogarci più seriamente di quanto abbiamo fatto sulle cause che l'hanno prodotto. Mi ha colpito molto quanto ho avuto modo di leggere ieri nel rapporto della commissione britannica, e non perché fossero cose per me sconosciute. Il Movimento pacifista le ha dette infatti tante volte nel corso di questi anni. Il punto è che le ha dette in maniera inascoltata, in maniera solitaria. Il punto è che quel Movimento, che denunciava come guerra e terrorismo si alimentassero l'una con l'altro, purtroppo è stato lasciato solo in tutti questi anni. Non c'è stata un'adeguata riflessione della politica rispetto a quanto soltanto nelle piazze, più che nelle Assemblee parlamentari, si aveva la forza di dire. Mi colpisce molto leggere che la commissione britannica dica con grande chiarezza non semplicemente che la guerra in Iraq del 2003 fu sbagliata, ma anche che quella guerra è stata una delle cause attraverso le quali si è formato il terrorismo fondamentalista. È un tema troppo serio per non diventare la riflessione principale che dovremmo svolgere in quest'Assemblea. Penso davvero che dobbiamo avere il coraggio di dire in queste ore così drammatiche che se vogliamo sconfiggere Daesh ci sono cose più efficaci, più utili e più importanti, dei bombardamenti. Dobbiamo, per esempio, avere la forza di dire che per sconfiggere Daesh bisogna fare di più per interrompere i flussi di finanziamento e di vendita di armi a quei Paesi che in questi anni hanno indirettamente o direttamente supportato Daesh. Dobbiamo avere la forza di dire che bisogna migliorare e strutturare maggiormente i nostri servizi di *intelligence*, per esempio aumentando il coordinamento sovranazionale. Dobbiamo però avere la forza di dire che noi sconfiggeremo Daesh se sapremo sconfiggerlo non solo militarmente, ma soprattutto culturalmente. L'ho detto mille volte in quest'Assemblea: è decisivo l'impegno dei Paesi islamici e l'impegno delle potenze sciite. Dobbiamo radicalmente ripensare ai rapporti, che pure ci sono stati in questi anni, con i principali esponenti del mondo sciita. Probabilmente anche su questo l'Occidente ha fatto degli errori nel giudicare quella minaccia addirittura ancora più grave di quella rappresentata dal mondo sunnita. Ebbene, bisogna mettere in campo una strategia politica. Credo, signor Ministro, che lei abbia ragione a dire che dobbiamo farlo unitariamente e che questo Parlamento debba farlo senza

Credo che se faremo questo, potremo ottemperare al grande sforzo che ho cercato di richiamare all'inizio di questo intervento: sconfiggere Daesh, senza modificare, nemmeno di un millimetro, la democrazia del nostro Paese Paese e la civiltà attorno alla quale abbiamo lavorato in questi anni. Signor Presidente, mi associo, a nome del mio Gruppo, alle parole del Ministro, che ho trovato ragionevoli, serie, come il suo appello all'unità, perché davanti a queste drammatiche vicende che riguardano i nostri connazionali non ci può essere spazio per pensieri in libertà. Questa vicenda del Bangladesh, drammatica, terribile, ci dimostra che nessuno è immune, né all'esterno né sul nostro territorio nazionale.

confidiamo nel Signore e naturalmente anche nelle Forze dell'ordine, ma teniamo presente che questa è una battaglia globale che non consente a nessuno di esprimere facili sicurezza. nessuno è al di sopra di ogni sospetto nel senso di poter essere tranquillo, né fuori dal territorio nazionale né in Italia. E fuori dal territorio nazionale non ci sono luoghi sicuri, perché quando si colpisce un luogo come un ristorante cambogiano a Parigi, Parigi, spiegatemi voi quale simbolismo può avere non una moschea, non una chiesa, ma un ristorante cambogiano a Parigi: nessuno. Ciò a dimostrazione che non ci sono zone e area in cui qualcuno può essere tranquillo. Questo è il mondo che noi stiamo vivendo e in cui dobbiamo abituarci a vivere. credo che dobbiamo fare una lotta senza quartiere non solo al Daesh, non solo all'ISIS, ma a tutti quei gruppi terroristici che si stanno stanno alleando in una lotta globale contro la civiltà. Non contro il mondo cristiano, non contro l'Occidente, guai a fare questo sbaglio: non facciamo lo sbaglio di pensare che ci sia la lotta ai ai cristiani o all'Occidente. Se facessimo una macabra contabilità dei caduti, ci accorgeremmo forse che in tutti questi attentati, pensate ai duecento morti di Baghdad, sono caduti più islamici che cristiani. Qui si cerca di minare le basi della coesistenza pacifica tra civiltà e religioni diverse. Probabilmente, se volessimo fare un grande favore e una grande cortesia a questi individui che impropriamente utilizzano l'Islam, dovremmo dire che c'è una guerra di civiltà e di religioni: avrebbero ottenuto il risultato che vogliono, che è esattamente quello che sollecitano con tutti questi atti dimostrativi. Lotta senza quartiere, dicevo, a tutti, dal Daesh ad Al Qaeda, da Boko Haram ad Al Shabaab. Prevenzione, repressione, mobilitazione e, consentitemi, sensibilizzazione.

riuscire a suscitare una capacità (molto sopita, diciamo la verità), di indignazione dell'opinione pubblica e di mobilitazione delle coscienze, anche dei nostri bambini e dei nostri giovani. È inutile spegnere loro la televisione davanti a questi fatti. È bene, invece, discutere con loro, e che anche il mondo scolastico si impegni a far maturare una consapevolezza comune. l'appello alla comunità islamica italiana: più energia, più forza, più coraggio nella condanna, meno timidezza.

che vengono da quei Paesi e che oggi tifano simbolicamente insieme a noi i colori della nostra nazionale di calcio. Noi dobbiamo chiedere ai rappresentanti ufficiali di questa comunità meno timidezza e dobbiamo lavorare perché ci sia una scuola italiana degli Imam, che possa in qualche modo formare chi deve a sua volta formare.

Benissimo, non apriamo alcuna moschea e apriamo invece centinaia di scantinati incontrollabili. Scusatemi, ma io preferisco ci sia una moschea piuttosto che centinaia di scantinati che nessuno è in grado di tenere sotto controllo, tantomeno le forze di polizia. Questo per dire che a volte, con la demagogia, si fa un gran danno. In conclusione, è stata demolita la tesi in base alla quale l'estrazione sociale difficile produce terroristi. D'altronde, solo chi non voleva vedere non ha visto in questi anni che il principe dei terroristi, Osama Bin Laden, nasce nei dintorni della famiglia reale saudita. E tutto il suo lavoro è finalizzato a cambiare l'equilibrio del mondo sunnita e dell'Arabia Saudita, contestando l'egemonia della monarchia regnante dei Saʿūd. per il principe dei terroristi, non avevamo certo bisogno di aspettare il Bangladesh per capire che esiste una questione drammatica. Che poi si vada a reclutare qualche disperato nelle *banlieue* parigine, questo senz'altro succede. Ma il fenomeno non può essere spiegato solo con la facile sociologia del bisogno perché, purtroppo, è ancora molto più complesso. simbolicamente, per dare questa prova di unità, caro senatore De Cristofaro, visto che lei ha appena citato Emmanuel, anche io voglio associarmi al suo ricordo a nome del nostro Gruppo parlamentare. Ricordiamo questo ragazzo, ragazzo, sfuggito a Boko Haram, che cercava serenità e tranquillità nella nostra Italia, che lavorava seriamente e aveva i suoi affetti vicino e che per difendere il decoro della sua fidanzata

un elemento simbolico fondamentale.

lei ha parlato di facili interpretazioni sociologiche, richiamate proprio ora anche dal presidente Casini, che in questa condizione, nell'attentato di Dacca, sarebbero state per una volta forse finalmente smentite.

è che nel suo discorso c'è stata una visione romantica della lotta al terrorismo, che non corrisponde alla realtà e neppure alle operazioni necessarie che il nostro Governo per primo dovrebbe mettere in campo per un'efficace lotta al terrorismo. Una visione romantica che ho notato soprattutto quando lei ha parlato dell'attrazione simbolica che hanno questi gruppi nei confronti di frange di popolazione povera o meno povera. No, signor Ministro, assolutamente no; non ci sarebbe attrazione simbolica che tenga se questi gruppi non ricevessero fiumi di denaro, o direttamente armamenti, dai governi occidentali o dai governi wahabiti. Ma quale attrazione simbolica avrebbero se fossero a mani nude? Lei nel suo discorso ha completamente dimenticato di ricordare che fiumi di denaro di provenienza "petrodollara" se mi posso permettere di utilizzare questo termine - arrivano a Daesh, agli altri gruppi e alle schegge impazzite che in questi giorni stanno mostrando come il contesto globale del fenomeno terroristico internazionale effettivamente stia cambiando, perché la minaccia è sì globale, signor Ministro, ma non dobbiamo dimenticare che nella lotta al terrorismo bisogna valutare anche le novità

mancano alcuni riferimenti ben precisi a come sia necessario isolare qualsiasi Governo che finanzi in maniera diretta o indiretta le formazioni terroristiche a ogni latitudine, dal Medio all'Estremo Oriente, dal Nord Africa al Centro Africa, all'Est europeo. In che maniera? Con una serie di sanzioni che il mio Gruppo ha sempre proposto e che devono essere avviate e sostenute in maniera seria e dura in sede nazionale ed europea. È vero che è necessaria una presa di posizione degli Stati islamici moderati; assolutamente sì, ma è altrettanto vero che è necessario un coordinamento delle forze di *intelligence*. D'accordo, ma questo è possibile e si può ottenere soltanto se abbandoniamo quella visione romantica, se pigiamo con forza

e con quei soldi si procura armi, tecnologia militare e non solo, da utilizzare contro i nostri cittadini.

lì sì ci sono centinaia di scantinati incontrollati dove i minori lavorano in condizioni di sfruttamento. Signor Ministro, ricordiamolo questo fatto, che non cancella il rispetto che abbiamo per le vittime italiane o qualsiasi altra vittima nell'attentato di Dacca. Non dobbiamo, però, dimenticare che la logica del capitale e del profitto in alcune situazioni porta porta nostri connazionali a esporsi. E sono quelli gli scantinati incontrollati che mi piace ricordare qui ora, caro presidente Casini, e non solo quelli dove si riuniscono, molto probabilmente spesso, gli islamici in Italia; anche quelli sono scantinati incontrollati. L'esortazione che le lascio, signor Ministro, e il contributo che voglio dare a nome del mio Gruppo è di non dimenticare mai il quadro di insieme e di non farlo con visioni di carattere assolutamente romantico. Badiamo ai fatti. Tagliamo i fondi a chi finanzia materialmente le formazioni terroristiche, perché sappiamo chi sono; lo sa la nostra *intelligence* e soprattutto lo sanno le *intelligence* dei Paesi nostri alleati.

polizia. Le lascio questa domanda, come riflessione ultima: chi mette bombe in casa degli attentatori? Qual è il disegno globale? Cosa sta accadendo nelle alleanze internazionali? Cosa spinge, soprattutto, soprattutto, una monarchia a mantenere ancora il prezzo del greggio a livelli così bassi per il proprio interesse, tanto da scatenare la fame e l'ingordigia delle compagnie internazionali? Dobbiamo stare attenti, signor Ministro, a come valutiamo la condizione e l'indifendibilità dei nostri connazionali. Non solo non dobbiamo fare in modo che siano indifendibili materialmente, ma dobbiamo fare in modo che essi siano difendibili da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista di un'azione corretta, continua, logica e coerente del nostro Governo e del suo Ministero, che in questo e in altri casi io e il mio Gruppo non abbiamo mai visto.

Signor Presidente, si chiamava Simona Monti, trentatré anni, aspettava un bambino. Eppure una persona come lei, che sarebbe stata risparmiata anche secondo il codice di guerra delle più efferate organizzazioni, è stata torturata, trucidata con un *machete*, insieme al bambino che aveva in grembo. Parlo di lei, una dei nove italiani assassinati nell'attacco terroristico di Dacca, per rimarcare a quale brutalità, a quale crudeltà, a quale assenza di umanità, arrivano i terroristi dell'ISIS, ubriacati dalla fede in un'interpretazione sbagliata e integralista della loro religione. Eppure non parliamo di persone inconsapevoli per ignoranza, visto che i terroristi in questione hanno frequentato le migliori scuole del Bangladesh. Né, tantomeno, il loro gesto è riconducibile a uno stato di povertà, a un sentimento di rancore verso una società in cui sono stati oggetto di privazioni e di sfruttamenti: tutt'altro, si tratta di persone che provengono da famiglie benestanti, inserite al meglio in quel mondo. Faccio questa premessa - e ringrazio il Governo per aver aderito alla richiesta avanzata dal mio Gruppo perché forse è arrivato il momento di squarciare quel velo di ipocrisia con cui il *politically correct* si rapporta con questi attentati che si consumano in decine e decine di località del globo. Per dire gli ultimi: un mese fa 49 persone sono state trucidate in una discoteca di Orlando; poco più di una settimana fa 45 persone assassinate nell'aeroporto di Istanbul e ora, appena tre giorni fa, quello che è accaduto a Baghdad. Appunto, l'ISIS ha trovato la ricetta giusta per colpire dove vuole, per globalizzare il terrore. E riesce a farlo in una maniera sicuramente più efficace e più spietata dei cugini, ormai demodé, di Al Qaida. L'ISIS si è trasformato in un *network*, in un'antenna che irradia odio su tutto il globo; in un esempio che, attraverso il *web*, raccoglie proseliti in ogni angolo del mondo: siano gruppi organizzati militarmente o lupi solitari, poco importa, tutto fa brodo. L'obiettivo che perseguono è quello di sempre: creare un'atmosfera di paura e di invincibilità. Non importa se i terroristi di Dacca fossero collegati più o meno direttamente con l'ISIS, o non lo fossero affatto, come sostengono le autorità di quel Paese. Il punto vero è che quel gruppo di disgraziati ne ha seguito l'esempio, ne ha messo in pratica i proclami, ha dato retta ai richiami della follia bestiale di Raqqa. Sono stati gli attori di quel copione studiato nei minimi particolari dalle menti abbiette dello Stato islamico in Siria e in Libia. Hanno applicato i dettami di quel *franchising* del terrore che è stato inventato a decine di migliaia di chilometri di distanza; dettami e principi che sono arrivati attraverso il *web*, attraverso i filmati da Istituto Luce che cantano le gesta dell'ISIS e che ne celebrano la potenza. se si vuole mettere fine a questi lutti, se non si vuole allungare l'elenco dei crimini efferati commessi sull'altare di una religione sbagliata, bisogna spegnere quell'antenna che irradia odio. C'è bisogno che l'ISIS perda quell'aureola di potenza, di impunità che si è costruita. Non bisogna accontentarsi dei successi militari, ma spazzare via in tempi brevi, sdradicare quel che ne resta in Iraq e in Siria, creando le premesse, se è possibile, di una grande collaborazione con gli Stati dell'Islam moderato e dando un maggior impulso a una grande coalizione internazionale in cui Stati Uniti e Russia collaborino davvero. Bisogna evitare che i terroristi sopravvivano più di quel che dovrebbero, complici le divisioni della comunità internazionale. L'obiettivo prioritario è porre fine a quest'esperienza devastante in cui il terrorismo si è fatto Stato: poi si potrà investire sulla cultura come dice il *Premier*; si potrà affrontare in maniera più efficace il problema dell'immigrazione, dei profughi di guerra; si potrà mettere ordine in quelle regioni maledette che non trovano pace; si potrà decidere il destino di Assad, si potrà dare spazio all'Islam moderato, che continua a contrapporsi con troppa timidezza al fanatismo, all'integralismo, alla violenza. Ma tutto passa - è inutile nasconderselo - per la fine dell'ISIS, perché in quel mondo conta, purtroppo, solo la forza. Altri discorsi sono una perdita di tempo e rimandano a un nuovo attentato, a un nuovo dramma. Si tratta di un obiettivo che va raggiunto subito, perché il tempo non è una variabile indifferente, perché più trascorrono i mesi e più assistiamo ai colpi di coda di quest'organizzazione, più l'odio attecchisce in qualche angolo remoto del mondo, a nostra insaputa. Questo massacro sta andando avanti da troppo tempo. Io non so se sia stato giusto spazzare via i regimi di Saddam o di Gheddafi. So solo, però, che la comunità internazionale ha la cattiva abitudine di aprire il vaso di Pandora e di lasciarlo marcire. In più mi colpisce un paradosso: per colpire i regimi di Saddam e di Gheddafi, che erano delle dittature ma rappresentavano Stati sovrani, la comunità internazionale in entrambi i casi fece guerre che durarono poco più di un mese. Poi ci sono stati i periodi di stabilizzazione, che ancora durano, ma in entrambi casi la guerra è durata poco più di trenta giorni grazie ad uno spiegamento di forze spettacolare. Invece, contro il terrorismo che si è fatto Stato, che conduce una guerra asimmetrica in tutto il mondo con le armi della paura, dell'odio, della tortura e degli omicidi di massa, l'iniziativa della comunità internazionale appare lenta e a volte indecisa e intanto i tentacoli di quel modo sbagliato di interpretare l'Islam si allungano verso altri territori, scrivono altre pagine di terrore. Dopo tanto aspettare forse è arrivato il momento che la comunità internazionale dica in tempi brevi davvero basta o almeno è questo il compito per il quale il Governo italiano si dovrebbe adoperare. prendo la parola a nome dei senatori e delle senatrici del Partito Democratico e in premessa intendo esprimere una condivisione senza riserve, nonché un vivissimo apprezzamento per la lucidità delle analisi e la passione dell'intervento del signor Ministro. Noi ci associamo anzitutto al lutto, al dolore per le vittime, alla sofferenza dei famigliari e dei loro cari, con un sentimento di orrore e insieme di medesimezza umana, di cristiana pietà e di laica commiserazione di fronte a una carneficina che è ultima di una lunga serie (a Parigi, a Bruxelles, ad Ankara, a Orlando, a Istanbul, a Bagdad); un crimine sanguinario ed efferato, una mattanza crudele perpetrata da fanatici mossi da una ideologia islamista radicale e fondamentalista. Siamo di fronte alla globalizzazione del terrore, a una nuova guerra asimmetrica, senza una linea del fronte, peraltro nel tempo di Internet e della mediatizzazione assoluta, Dopo le recenti sconfitte subite da Daesh nella terra di Sirak, la lotta si estende a Sud dell'Oriente. Non è una semplice esportazione, ma pure è la presenza di nuove insorgenze. Ebbene, a nostro avviso, la risposta va perseguita non facendoci travolgere dal cumulo delle emozioni e dei risentimenti, pure legittimi e comprensibili, o da spirito di vendetta, ma affidandoci alle mosse della ragione che persegue la giustizia.

parla di un Islam radicalizzato, vale a dire di una linea di teologia politica entro la quale la teologia è il mezzo e la politica è il fine. È questa l'ideologia di ceti intellettuali e borghesi urbani,

per ISIS e Daesh? È certamente il crociato e l'infedele, ma pure l'apostata, come apostata è Hossein Faraaz, che cade per difendere donne cristiane, donne e uomini musulmani. Il nemico è l'intera civiltà umana. C'è pure - Roy ce lo insegna - un radicalismo in declinazione islamista che si regge su basi sociali diffuse. A questo proposito divergo dall'interpretazione di colleghi di cui ho largamente condiviso l'impostazione.

La linea di congiunzione tra queste due linee sta esattamente nella politica del terrore che non ha barriere territoriali e sociali e che si intreccia a conflitti regionali, a contrapposizioni storiche, alla guerra civile intramusulmana, tra sunniti e sciiti, a responsabilità di scelte sbagliate dell'Occidente. Ci sono pure linee di frattura e di divisione tra l'Islam spirituale e religioso e l'Islam politico, a loro volta lacerati tra riformisti e radicali, tra modernizzazione dell'Islam

Ebbene, quali possono essere le risposte? La mia condivisione con il Ministro giunge quasi a una sovrapposizione. Innanzitutto dobbiamo restare noi stessi e promuovere e tutelare i nostri valori e la nostra identità,

nel contributo che possiamo dare, insieme agli amici islamici, alla nascita e allo sviluppo di un Islam europeo, di un Islam che possa condividere i valori, i principi, le pratiche della cultura civile La seconda risposta sta nella politica. Dobbiamo individuare con precisione il nemico e distinguere amici e nemici. Dobbiamo ricompattare il fronte atlantico, dialogare con la Russia di Putin, far capire chiaramente a taluni, alle monarchie e alle petromonarchie che il tempo del doppio gioco è scaduto, che non c'è un mondo o una terra di mezzo di fronte a Daesh e all'ISIS. da perseguire, noi dobbiamo potenziare le nostre strutture di sicurezza, l'*intelligence*, la polizia, rafforzare i meccanismi di prevenzione, reagire con fermezza e repressione Non dobbiamo, da democratici, avere paura della parola «repressione». *(Applausi del senatore Sonego)*. Dobbiamo infliggere, con azioni mirate, colpi volti a minare l'aura di invincibilità, l'attrazione simbolica, le fonti di finanziamento di Daesh. Infine, dobbiamo irrobustire e consolidare l'unità della nostra Nazione, di tutte le forze democratiche. Il che significa anche resistenza - per a quella tentazione fuorviante che unifica e identifica musulmano e terrorista, rifugiato e jihadista. Questa è una prospettiva distorcente, perché si tratta di non essere nemici a noi stessi, consentendo così ai nostri morti, ai nostri martiri, alle vittime innocenti - testimoni di un'Italia laboriosa e intraprendente - di poter riposare in pace.

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per ricordare in quest'Aula l'assassino di Emmanuel Chidi, di trentasei anni, nigeriano, richiedente asilo, ucciso a Fermo da una vile e infame aggressione razzista. E voglio ricordare questo assassinio in questa

per cui molto di frequente si lasciano correre frasi terribili, che poi sedimentano e crescono. L'episodio di Fermo di ieri non è isolato, se solo stiamo alla cronaca recente, che parla di aggressioni a Parma, a Firenze. Voglio ricordare la vicenda di Emmanuel e della sua compagna, Chinyery,

vittime su vittime in un crescendo sanguinario. Emmanuel e Chinyery hanno attraversato il Niger, la Libia e poi, su un gommone, il mare di Sicilia. Per la durezza di un viaggio terribile - lo sappiamo - Chinyery, incinta, ha perduto il suo bambino, una volta arrivati a Lampedusa. Da Lampedusa si sono trasferiti poi a Fermo, dove hanno cercato innanzi tutto di ricostruire una nuova vita, in attesa dello *status* di rifugiati. Accolti dalla comunità di Capodarco, sono stati sposati illegittimamente - in un atto quasi di disobbedienza civile - da don Vinicio Albanesi il 6 gennaio di quest'anno nella chiesa di San Marco di Fermo. La nuova vita è stata interrotta drammaticamente, con una modalità bestiale, due pomeriggi fa, quando Emmanuel e Chinyery stavano attraversando una delle vie centrali della città, a pochi metri dalla piazza principale, e sono stati apostrofati duramente da due nostri concittadini, uno dei quali ha ripetutamente detto a Chinyery di essere una scimmia. Di fronte alle proteste di Emmanuel, la risposta è stata un'aggressione senza tregua: con un palo divelto Emmanuel è stato massacrato, colpito ripetutamente anche dopo aver perso i sensi, la violenza si è abbattuta anche sulla sua compagna Chinyery. Dopo molte ore di coma, Emmanuel ieri è morto nell'ospedale di Fermo. Signora Presidente, penso

il linguaggio dell'odio, della paura, dello scherno e della mancanza di rispetto. Quanti sono anche i casi di femminicidio nel nostro Paese? Quanti i casi di aggressione nei confronti degli omosessuali nel nostro Paese? Quanti i casi di aggressione razzista nel nostro Paese? Non possiamo operare alcuna rimozione

Signora Presidente, non so cosa sia successo ieri. Poi impareremo e approfondiremo l'accaduto.

Senatore Giovanardi, non ha la parola sull'ordine dei lavori.

Il dibattito che è seguito alle dichiarazioni del ministro Gentiloni Silveri ha dimostrato che il Paese è compatto nel difendere i propri valori. Poi è stato ricordato un gesto, il quale non ci sono parole, un gesto di vigliaccheria, che ha portato a morire una persona;

che apparteniamo ad uno Stato democratico, che rispetta gli uomini e le donne di qualsiasi razza, di qualsiasi religione e di qualsiasi credenza. *(Applausi

forse non era opportuna. Ma lei è la Presidente, in questo momento e quindi rispetto la sua decisione. Visto e considerato che si è iniziato a parlare di quanto è successo, io io dico, senatore Giovanardi, che so quello che è successo ieri, perché l'ho appreso dagli organi di informazione: un assassino ha ucciso una persona. Un assassino - ripeto

assassino è bianco, ma poteva anche essere nero, rosso, giallo, verde; poteva arrivare da Marte, da Fermo, da Pavia o da chissà quale altro posto dell'universo. È un assassino. Di conseguenza, quello che chiediamo in quest'Aula e che continuiamo a chiedere da mesi, forse da anni, è che ci siano tre parole:

tanto sa benissimo che non succede niente e non gli succede niente. Questo non è solamente l'episodio di razzismo che deve essere condannato, perché le persone si giudicano non per il colore della pelle, ma per quello che hanno dentro, per quello che portano e per quello che sanno dire e fare.

Finalmente possiamo dire quanto gli italiani sono razzisti e cattivi. In queste ore gli organi di informazione finalmente hanno trovato l'assassino

Nessuno in quest'Aula ha mai speso una parola strumentalizzare! PRESIDENTE. Lei continui a parlare e io faccio il mio lavoro. Ho già richiamato i colleghi alla mia sinistra perché le consentano di parlare. Continui il suo intervento.

il biglietto del treno! E, allora, prima di riempirvi la bocca, pensate a quello che sta succedendo nel nostro Paese per colpa vostra!

il reato di tortura è necessario. Ahimè, non è scontato ribadirlo e sottolinearlo. Perché, cari colleghi? È semplice: manca nel nostro codice. In tante legislature si è provato ad inserire il reato di tortura, tutti i tentativi sono andati falliti, legislatura dopo legislatura. Cari colleghi, abbiamo tutti insieme la responsabilità di non mancare a questo importante appuntamento. Il reato di tortura è necessario perché utile a colpire particolari condotte. Colleghi, il nostro codice copre la minaccia, la violenza, le lesioni, l'omicidio condotte gravi - con delle pene severe. Ma siamo sprovvisti di una norma in grado di colpire il tipico reato di tortura che, rispetto a quei gravissimi comportamenti, ha un disvalore accentuato e particolare che merita l'intervento del legislatore. colleghi, il reato di tortura è necessario perché risponde alla scelta di aderire alle convenzioni internazionali, innanzitutto alla Convenzione di New York del 10 dicembre 1984, con cui in modo solenne si chiede a tutti gli Stati di prevedere il reato di tortura, richiamandosi all'articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

si definirono le istituzioni e le procedure che gli Stati membri debbono adottare per monitorare i casi di violazione di diritti umani e di tortura.

ad avere un comportamento coerente, in grado di poter dire che il nostro Paese ha tutte le carte in regola.

che dà conto del lavoro legislativo a cui tutti siamo chiamati al di là della funzione che abbiamo, sia di maggioranza che di opposizione. Ieri, in discussione generale sono emerse le caratteristiche del reato di tortura. Ho apprezzato moltissimo l'intervento del senatore Manconi, Presidente della Commissione a tutela dei diritti umani qui al Senato, ha spiegato bene le caratteristiche del reato di tortura: avvilisce la persona, ne degrada la condizione umana, ferisce e annienta la sua dignità, produce sofferenze inenarrabili e ha diverse finalità punitive,

dare il nostro consenso all'introduzione del reato di tortura. Noi, come Partito Democratico, ci siamo spesi perché fosse raggiunto un equilibrio tra l'attenzione alla tutela dei diritti umani, che a gran voce ci viene richiesta anche in queste ore da tante associazioni, da tanti esperti e cittadini, e la necessità

di inibire l'uso democratico della forza. Niente paura. Niente giudizi. Niente disdoro. Al contrario, mettere al loro servizio uno strumento in più per fare in modo che anche il loro importante lavoro possa scorrere lungo i binari della massima correttezza e della massima tutela dei diritti inviolabili delle persone. Penso che questo equilibrio sia stato raggiunto. Ecco perché invitiamo tutta l'Assemblea a votare questo provvedimento. Si è fatta la scelta di concepire la struttura del reato come reato comune. Anche questa è stata una scelta equilibrata, perché la tortura può essere consumata da diversi soggetti. Sulla pelle del nostro Paese abbiamo sperimentato questa maturazione e le scelte che adesso ci apprestiamo a fare. Pensate alle mafie, alle cosiddette camere della morte, dove delle persone sono stato portate e hanno subito degli orrori sulla loro psiche e sul loro corpo. Alla fine, molti di questi sono stati anche sciolti nell'acido. Pensiamo al piccolo Di Matteo. Pensiamo anche ad altre forme di criminalità che abbiamo conosciuto. Pensiamo ai casi dei quali sono stati proiettati anche dei filmati, come alcune case di riposo e alcuni asili nido. Ecco perché abbiamo fatto la scelta di considerarlo reato comune. Naturalmente non ci siamo sottratti, così come le convenzioni internazionali ci richiedono, a prevedere delle aggravanti per il pubblico ufficiale e per l'incaricato di pubblico servizio. È un equilibrio, a mio avviso positivo e fecondo, che ci può mettere nelle condizioni di votare e licenziare questo provvedimento. Ecco perché, cari colleghi, signora Presidente, in questa legislatura possiamo scrivere una pagina positiva ed essere orgogliosi di un Parlamento che ha fatto delle scelte, ha coperto un limite e ha saputo dare una bella autorevolezza in questo particolare momento al nostro Paese.

Presidente, mi permetto di replicare, data la delicatezza del tema e la necessità di fare chiarezza su questioni che possono avere una apparente fondatezza. Per questa ragione, l'Assemblea deve riflettere sui punti che mi permetterò di esporre da qui a qualche momento.

in una sorta di doppia opposizione al testo. Per un verso, si dice che il delitto di tortura, per come noi lo abbiamo pensato e scritto, restringerebbe troppo l'area della punibilità. In altri termini, si pretenderebbe una fattispecie più dura e un ampliamento del cerchio della punibilità. Per altro verso, si dice che con questa norma troppa dilatata (ecco perché parlavo di critiche di segno del tutto opposto) noi mettiamo le forze di polizia in una condizione di difficoltà. Proprio l'estrema divaricazione delle due critiche è dimostrativa della natura equilibrata del testo che già

sufficiente, ho in un certo senso classificato per gruppi e categorie generali gli emendamenti proposti e su questi darò una risposta, premettendo però una avvertimento importante: il diritto non è una categoria ideologizzabile non è una categoria dello spirito. Una norma si inserisce in un sistema e sarebbe del tutto incongruo scrivere una norma che non tenesse conto del sistema dentro il quale è destinata a operare. Si dice che, per restringere il campo di applicazione della norma, avremmo dovuto introdurre un dolo intenzionale, ovvero l'avverbio «volontariamente»: è una componente che ricorre con una certa frequenza negli emendamenti proposti. Il «volontariamente» è certamente superfluo; tutti i delitti sono dolosi e quindi sono volontari. Non c'è dubbio e sarebbe - direi - un errore tecnico piuttosto imbarazzante. Quanto alla scelta dell'«intenzionalmente» ora qui dico una cosa, cosa, peraltro ovvia: ci sono determinati delitti che, per la loro struttura oggettiva, implicano condotte che sono tipicamente intenzionali, direi fortemente caratterizzate sul versante del dolo. È pensabile che chi operi violenze reiterate e minacce gravi a una persona privata della libertà personale, che cagioni quei risultati, lo faccia per colpa o lo faccia distrattamente, per imprudenza, imperizia o negligenza? È chiaro che l'introduzione di qualificazioni della componente soggettiva è del tutto superflua, direi che si tratterebbe di un vistoso errore. Si sottolinea poi la necessità di introdurre varie cause di non punibilità: si dice «uso legittimo delle armi», necessità di fare uso non soltanto di armi, ma di ogni altro mezzo di coazione al fine di respingere una violenza o di vincere una resistenza. queste sono componenti di storiche scriminanti che stanno nel nostro sistema penale. È chiaro che queste scriminanti non debbono e non possono essere inserite all'interno della norma, in quanto operano autonomamente in via del tutto automatica. se il pubblico ufficiale avrà agito nell'esercizio, appunto, di un obbligo giuridico che caratterizza l'esercizio delle sue funzioni nell'adempimento di ordini legittimi e peraltro non sindacabili (non entro troppo nel dettaglio della questione), questo pubblico ufficiale non sarà punibile. Il legislatore inserisce nella parte generale tutta una serie di istituti che automaticamente e senza alcuna necessità di richiamo si applicano alla parte speciale. Sostanzialmente si dice (ma questa è una critica opposta): "Voi avete scritto «violenze o minacce» peraltro «reiterate»; qui dovrebbe bastare una sola violenza o una sola minaccia". Questa scelta non la si può con assoluta certezza percorrere, perché se questo avessimo fatto, non avremmo potuto spiegare la differenza sanzionatoria che costituisce l'intervallo che separa una violenza privata o una minaccia

fosse stata ritenuta sufficiente a classificare il delitto di tortura, altro non avremmo fatto che sovrapporlo a delitti preesistenti: la minaccia nelle sue forme non aggravate o aggravate, la violenza privata e altri reati che sono contestabili. Qui dobbiamo avere la convinzione, che costituisce d'altronde il risultato di una banale constatazione, che quando parliamo di tortura interveniamo su di un terreno rispetto al quale le norme già esistono, norme diverse che vanno contestate in concorso. Andava tipicizzata la forma del delitto di tortura, ma certamente non la si poteva tipicizzare costruendola su norme già esistenti. Poi, ovviamente, la giurisprudenza e la dottrina avrebbero avuto gioco facilissimo nel dire che il Parlamento è disattento rispetto al sistema e che non si coordina culturalmente per come dobbiamo al contrario fare. Poi si dice che si dovrebbe inserire «aver praticato sevizie» o «agito con crudeltà». La crudeltà c'è già, quindi direi che vi è una certa distrazione sul testo: le sevizie sono implicate dalle violenze le norme non possono scontare delle superfetazioni, delle ripetizioni, che ne complicano il processo di applicazione. Si critica, poi, il «verificabile trauma psichico». Devo fare un passo indietro: non potevamo trascurare quelle lesioni di natura psichica, quella malattia psichica - per usare un termine più confacente al linguaggio, perché lesione significa, appunto, malattia che avesse un contenuto di natura psichica. Se a seguito di torture, di qualsivoglia natura, taluno avesse subìto un trauma psichico ma non una lesione personale sarebbe stata dispari una stata dispari una disposizione che avesse, al contrario, previsto la punibilità soltanto per una malattia di natura fisica. È chiaro però - e, in un certo senso, la norma è accorta ma, potrei dire,

la psichiatria moderna ha strumenti indiscutibili, condivisi a livello mondiale, di verifica dei traumi psichici. Non è che, in questo caso, stiamo pensando alle categorie dell'impossibile o dell'astrazione. Il *Thermal Rorschach* e l'MMPI, tanto per fare alcuni riferimenti banali, sono strumenti collaudati dalla psichiatria mondiale per verificare il trauma. un buon giudice - ma direi, ogni giudice - dinanzi alla dichiarazione di aver subìto un trauma psichico ricorre inevitabilmente a una verifica, che si espleta attraverso il conferimento di un incarico psichiatrico. Ho visto anche contestare quella pena che giunge purtroppo - e sottolineo il purtroppo, con un doppio significato: purtroppo per la vittima, principalmente, ma purtroppo anche per l'imputato, che ne subisce le conseguenze della tortura alla quale consegua la morte, che è punita con la pena di trent'anni di reclusione.

le quali ovviamente andavano trattate alla stessa maniera. Abbiamo costruito, credo, una norma equilibrata sul divieto di respingimenti, espulsioni, estradizioni, allorquando vi sia il

Questa individualizzazione della verifica del rischio di tortura è, ciò nonostante, mediata da una valutazione ulteriore, ma accessoria, secondaria, in virtù della quale si dice che si tiene conto delle violazioni sistematiche dei diritti umani, nel caso in cui quel soggetto fosse respinto verso un Paese in cui i diritti umani sono sistematicamente violati.

(sia quella del pubblico ufficiale, sia quella dell'incaricato del pubblico servizio) non sono ovviamente riscontrabili. È chiaro che abbiamo dato maggiore risalto punitivo alla tortura compiuta da soggetti pubblicistici, perché si tratta di soggetti rispetto ai quali è giusto pretendere una maggiore tassatività di fedeltà rispetto agli obblighi che incombono sulle loro funzioni, ma era impensabile lasciare fuori le tante ipotesi riconducibili a questo testo che avvengono in contesti privati. La illustrazione e la replica agli emendamenti, ma anche l'espressione dei pareri che il relatore Buemi farà daranno conto peraltro di aperture che abbiamo ritenuto doveroso operare per la qualità degli emendamenti e per la bontà delle argomentazioni che stavano alla loro base; di talché il testo non è caratterizzato da una sorta di resistenza a tutti costi da parte di chi lo ha scritto, nel senso che si è ritenuto di non accettare i tanti giusti fondati consigli; ripeto che il senatore Buemi ne darà conto, perché noi alcune indicazioni importanti abbiamo ritenuto di doverle accogliere. È per questa ragione che mi permetto per la terza volta - e mi scuso per la ripetizione - di affermare che questo è davvero un testo equilibrato.

dal punto di vista della necessità di introdurre nel nostro ordinamento un reato che non era previsto, sia per il contesto che esso ha prodotto. Vorrei altresì ricordare che il presente è uno degli obblighi che il nostro Stato ha dovuto assolvere nel corso degli anni caso vorrei dare puntuale conto di ciò che il nostro Paese ha realizzato nei termini di prevenzione della tortura e di adesione ad altre modalità che hanno inteso Non si tratta quindi semplicemente di un adeguamento di carattere codicistico, ma del completamento di un percorso che, come è stato autorevolmente ricordato in Si tratta quindi - e sono risuonate parole importanti proprio stamattina nel corso dei dibattiti precedenti - di porre l'attenzione massima a ciò che prevede e prescrive la nostra Costituzione in termini di protezione dei diritti umani e di divieto della tortura al pari di ogni trattamento crudele, disumano e degradante. In questo senso vorrei ricordare che il divieto è previsto sia nella Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'articolo 3, sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all'articolo 7. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 poneva il divieto, pur con delle limitazioni di non poco conto (morale, di ordine pubblico) a questa fattispecie. Infine, la più volte richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, è in vigore dal 26 giugno 1987. Il richiamo delle date non vi appaia superfluo o semplicemente nozionistico perché vorrei far comprendere, dal nostro punto di vista, come questa discussione e l'adozione anche di questa Convenzione siano state prodotte in un contesto - la metà degli anni Ottanta - nel quale c'erano ancora molte dittature a livello internazionale. Era da poco terminato il regime della guerra sporca della dittatura argentina; erano in vigore in molti Paesi, anche in Europa, dei regimi di carattere dittatoriale e c'era l'*apartheid* in Sudafrica. Il fatto che sia stata ratificata dopo tre anni

Il fatto che nel nostro Paese con un processo legislativo si sia portato alla ratifica il 3 novembre 1988 e poi alla vera adozione l'11 febbraio 1989, quando fu poi consegnata alle Nazioni Unite questa autorizzazione, ritengo debba farci riflettere non solo sui ritardi odierni, ma anche sulla difficoltà che ha comportato l'adozione di questa norma. È importante richiamare anche in maniera puntuale cosa prevede, nell'articolo 1, la nozione di tortura, in modo che possa esserci utile nel nostro compito di legiferare.

e minaccia. La Convenzione rappresenta, per quanto ci riguarda, un punto fondante della civiltà giuridica nostra e dell'intero consesso dei Paesi civili. civili. L'idea che si possa assumere quello che è già presente all'interno del nostro codice come sufficiente a punire il reato di tortura deve essere rimossa, a nostro giudizio, da una discussione che altrimenti apparirebbe fuorviante. È per questo motivo che, nonostante il nostro Paese abbia adempiuto agli obblighi di sottoporsi ai periodici controlli dei comitati e delle agenzie che presiedono al controllo delle attività, anche nell'esercizio delle funzioni pubbliche, che prevedano la possibilità di il nucleo della Convenzione ci impone la necessità di legiferare. In particolare, gli articoli 1 e 4, in combinato disposto, propongono questo tipo d'iniziativa.

Il mio compito qui è indicare il nucleo fondamentale intorno al quale si costruisce questa ipotesi di reato. quindi, è quello di dare conto anche di un'evoluzione, non solo normativa ma anche di convenzioni, che è stata poi oggetto di una successiva intenzione da parte delle Nazioni Unite. cosiddetto OPCAT, il Protocollo opzionale dell'ONU alla Convenzione contro la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumano e degradante, che è del 2002, è stata autorizzata dal Parlamento - pensate un po' - con la legge n. 195 del 2012, con un ritardo di dieci anni, con relativo ordine di esecuzione. Il Protocollo prevede il meccanismo di prevenzione nazionale, che doveva essere designato o creato entro un anno alla data di entrata in vigore. È evidente che l'adozione del Protocollo opzionale non ha mutato, però, il contesto legislativo entro il quale ci siamo mossi. mossi. Tale Protocollo opzionale rappresenta una valida sintesi del contributo che ai lavori preparatori hanno dato non solo organismi di carattere istituzionale e governativo, ma anche organizzazioni non governative. per dare il senso che su questo tema e sulla sensibilità nella protezione dei diritti umani ci debba essere sempre un proficuo e articolato confronto con quelle organizzazioni della società civile e non solo con i termini giurisdizionali, che tanto hanno contribuito a far crescere una consapevolezza intorno a questi temi. È per questo motivo - lo vorrei ricordare - che, anche sulla base di precisi e sistematici richiami della giurisdizione internazionale, è stato istituito nel nostro Paese il Garante nazionale dei detenuti,

in cui la tortura è proibita dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 nonché dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, del 1987, ha subito un ulteriore implementazione da due protocolli nel 1993. L'Italia è parte di tutti questi strumenti e l'organo di controllo della Convenzione europea per la prevenzione della tortura, il CPT, agisce con sistematiche missioni anche di controllo all'interno del nostro Paese. Si tratta, quindi, di evidenziare le lacune normative, che qui vengono coperte dall'introduzione specifica del reato, in modo tale che vi sia una fattispecie incriminatrice specifica. poi questa abbia - lasciatemi dire - un'estensione anche al regime privato a me sembra un rafforzamento di quelle garanzie che rappresentano anche gli obblighi costituzionali ai quali noi dobbiamo rispondere. Fino ad oggi mancava la determinazione della pena; con questa legge si istituisce, e dev'essere necessariamente stabilita, una relazione in modo tale che possano essere tipizzati i reati che vengono condannati. Analogo discorso - e forse tra i più importanti, anche per il richiamo che è venuto da sentenze della Cassazione e della Corte EDU - riguarda la prescrizione del reato, che fino ad oggi, essendo rapportato a fattispecie criminose previste esplicitamente dal legislatore, risultava troppo breve rispetto a quelle che vengono previste come lesioni e lesioni e abuso d'ufficio, agli articoli 608, 572 e 582 del codice penale. In questo senso, l'introduzione del reato sana anche questo aspetto, consentendo che la prescrizione non intervenga su una fattispecie fattispecie criminosa tanto odiosa. Questo è tanto importante quanto lo è il richiamo alla non estradizione o espulsione verso i Paesi dove i soggetti siano a rischio di tortura. Anche questo rappresenta non solo un'ambizione, ma anche un convincimento profondo del nostro Governo relativamente a quali siano i suoi obblighi nel difendere quei diritti di civiltà che rappresentano la materia viva della Costituzione materiale del nostro Paese rispetto alla sua presenza nel consesso internazionale. vorrei ricordare anche quali sono stati gli impegni precisi a seguito di sentenze, come quella del cosiddetto

le violenze in causa erano state perseguite come lesioni personali, semplici o aggravate, in relazione alle quali, in applicazione dell'articolo 157 del codice penale, era intervenuta la prescrizione nel corso del procedimento.

all'articolo 3, in tema di divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. A tal proposito, vorrei citare il testo della sentenza della Corte europea di Strasburgo: «La Corte ritiene necessario che l'ordinamento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e a impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte».

anche sottolineare che l'ampliamento dell'applicazione della norma sul piano soggettivo e su quello oggettivo nel caso dei funzionari rappresenta una più puntuale descrizione della fattispecie incriminatoria. È per questo motivo che è stata introdotta un'aggravante specifica per quanto riguarda gli agenti e gli ufficiali di polizia,

è importante dare il senso di una piena capacità di intervento del nostro Governo e del nostro Stato nel perseguire questo reato.

condizione di immunità che, all'interno del nostro ordinamento, può essere considerata valida per opporsi all'incriminazione per il reato di tortura. è importante anche nel caso in cui ci si trovi di fronte a contesti nei quali sono coinvolti cittadini stranieri, dotati tanto di immunità funzionale quanto di quella diplomatica. È questo il senso dell'introduzione di un reato di tortura. C'è la nostra volontà di colmare le lacune del diritto interno e di costituire una norma di chiusura nell'ordinamento, in relazione alle garanzie di tutti i cittadini.

ad ulteriore corredo di quanto ci riguarda in caso di obbligo internazionale, ci dice che bisogna ragionare sui limiti della forza e sulle prerogative dell'esercizio della forza, in modo tale che siano tutelate le funzioni pubbliche e siano tutelati i diritti inviolabili dei cittadini. Sono vicende e sono diritti che devono essere garantiti, in modo tale che non vi possa essere alcuna omissione

da definire un quadro più esaustivo, più completo e più funzionale al perseguimento degli obblighi costituzionali e dei precisi doveri politici e civili che quest'Aula e questo Parlamento si propongono.

Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi del relatore e del Governo, c'è ancora più incertezza in merito a questo provvedimento e a quello che sarà poi il riverbero reale che avrà sui tutori dell'ordine. Per tale ragione, ai sensi dell'articolo

considerare se le cose dette vengono fatte perché si ignorano i fatti o per malafede. Ieri il senatore Cappelletti ha indicato come caso di tortura il caso di Federico Aldrovandi, dicendo che non c'è dubbio che vi sia stata tortura. Ho portato qui la sentenza, che rispetto e che vado

la perizia di parte è arrivata a conclusioni diverse e la sentenza dice: «Non è ragionevolmente immaginabile che quattro agenti di esperienza come gli odierni imputati non fossero al corrente del rischio di una asfissia da restrizione nella situazione nella quale si sono trovati ad operare,

la posizione in cui l'hanno tenuto per imperizia ha determinato la condanna per omicidio colposo. Noi ci dobbiamo allora mettere d'accordo su cosa succede in casi come questi, colposi e non dolosi.

ad esempio, al turbamento psichico accertato. Sostiene giustamente il relatore che saranno poi i periti a stabilire se questo turbamento psichico ci sia stato o no. Sì, ma nel frattempo l'accusa è quella di tortura, che è un reato che, nei casi citati dal collega Cappelletti,

Secondo questa interpretazione, quando i carabinieri davanti a Palazzo Chigi lo hanno immobilizzato, tenendolo per terra prono e gli hanno messo le manette dietro la schiena, se fosse intervenuto l'infarto di Preiti, come in quel caso, quei Carabinieri, se si se si definisce tortura questo tipo di atteggiamento, sarebbero finiti all'ergastolo. Ebbene, capisco la preoccupazione dei cittadini e delle Forze dell'ordine. Un ripensamento per scrivere meglio queste norme è necessario perché abbiamo visto, sentito sono state dette esplicitamente cose che sono evidentemente un pregiudizio nei confronti delle Forze dell'ordine e non una serena valutazione dei rischi, dei pericoli e della necessità di colpire il dolo. I fratelli Savi è giusto che siano in galera e all'ergastolo sette volte per quello che hanno fatto e così carabinieri e poliziotti infedeli che si macchiano di delitti dolosi. Quando però il collega Parisi ha ricordato che un pubblico ministero ha detto che il caso Cucchi è come il caso Regeni, c'è da indignarsi. Tutti dovrebbero indignarsi con paragoni di questo tipo rispetto ad una tortura bestiale di cui Regeni è stato vittima ed è stato ucciso e i casi di cui stiamo parlando. Certo, se si confondono i due piani c'è da essere preoccupati come cittadini e come Forze dell'ordine.

all'esame degli articoli, anche a partire dalle motivazioni che sono state addotte per questa richiesta. Non spetta al Parlamento stabilire in quale caso specifico ci sia stata, ci sarà tortura oppure no. una cosa che spetta alla magistratura, che lo farà, come lo ha già fatto in sede nazionale come in sede europea, a fronte di tristi e note vicende accadute nel nostro Paese. A noi spetta varare una norma generale senza entrare nel merito dei singoli fatti di cronaca. La stagione delle leggi *ad personam* in questo Paese

e non si tiri in ballo la credibilità delle Forze dell'ordine, che è una cosa che a noi sta molto a cuore ed è proprio per fornire alle Forze dell'ordine, che nella loro quasi totalità hanno atteggiamento di grande correttezza e da servitori dello Stato, uno strumento ulteriore di garanzia uno strumento ulteriore di garanzia della trasparenza e della legittimità della loro azione, che noi oggi andiamo a proporre l'approvazione di questo

per poter avere la possibilità di discutere ulteriormente queste norme. La Commissione ha fatto un lavoro sicuramente molto positivo, pertanto

il pericolo è il seguente: chiunque (e certamente noi che siamo garantisti dei diritti del cittadino nei confronti di qualunque abuso da parte dello Stato e di persone che a nome dello Stato devono svolgere determinati compiti) ritiene condannabile sotto ogni punto di vista nel modo più grave i i maltrattamenti gravi e la tortura nei confronti di persone sottoposte a restrizioni della loro libertà. E vanno intraprese le misure necessarie a fare sì che questo comportamento venga punito. Ecco perché vi è il ritiro dell'emendamento 1.200 soppressivo dell'articolo che sarebbe soppressivo dell'intero provvedimento. Tuttavia bisogna evitare

si è tornati a un testo simile a quello originariamente approvato dal Senato, che dunque si rivolge a tutti. Ricordiamo che con il testo approvato da quella che molti vorrebbero fosse l'unica Camera, Camera, le più efferate, sistematiche torture, che da tutti potrebbero essere riconosciute come torture gravissime, non sarebbero state colpite da questo reato purché non si fosse trattato di pubblico ufficiale.

alle Forze dell'ordine. Questa è una stortura che si è evitata, ma va ricordato che le Forze dell'ordine purtroppo non hanno a che fare sempre con dei gentiluomini, poiché spesso devono trattare con delinquenti - e la cosa non dovrebbe sorprendere - che conoscono benissimo gli strumenti attraverso i quali tentare artificiosamente di accusare chi è addetto alla loro difficile sorveglianza di reati gravi, che con questo provvedimento diventeranno ancora più gravi. Ecco perché ci sono vari emendamenti, che poi verranno evidenziati durante la discussione, in cui in cui si specifica, ad esempio, che vengono esentate in ogni caso le sofferenze che possono essere inflitte durante l'esercizio legittimo e nel rispetto della legge della forza pubblica nelle manifestazioni di ordine pubblico. Cosa ben diversa è

non si deve poter essere perseguiti. Nell'eseguire l'ordine di sgomberare dei manifestanti violenti, infatti, può capitare di colpire, anche ripetutamente, una persona. Dobbiamo evitare che si confonda chi svolge il proprio dovere con chi, abusando

Su argomenti così delicati, io trovo sia indice di poca sensibilità dividersi su posizioni da stadio, facendo il tifo per una posizione piuttosto che per un'altra. E ho apprezzato molto l'intervento del Presidente della Commissione giustizia, proprio nel tentativo di trovare equilibrio tra le diverse istanze che sono alla base di questo provvedimento. Prendendo spunto proprio dall'intervento del Presidente della Commissione giustizia,

noi riteniamo che queste norme non siano così tautologiche. L'elemento che riguarda molti degli emendamenti che abbiamo presentato, come quello sulla questione della volontarietà da aggiungere all'azione della crudeltà, viene molto spesso richiamato (e credo sia questo il motivo fondamentale) soprattutto dalla Convenzione

questo elemento, il fatto che la volontarietà è quell'elemento distintivo attraverso il quale nella viene evidenziato il dolo. Dunque il richiamo in questi emendamenti per noi è fondamentale anche per l'approvazione finale del provvedimento.

1.262 si riferisce all'articolo 613-*ter*: «Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura». L'emendamento, molto semplicemente, mira ad aumentare la pena edittale, prevista nel provvedimento

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Ora il reato di istigazione a delinquere, previsto dal codice penale all'articolo 414, per qualsiasi tipo di delitto prevede una pena da uno a a cinque anni di reclusione. Risulta un po' difficile comprendere perché chi istiga a commettere un delitto, quale può essere qualsiasi altro delitto, punito con pene anche inferiori a quelle che prevediamo per la tortura (un furto, una rapina, un qualsiasi delitto), debba essere soggetto a una sanzione minima di un anno, mentre il pubblico ufficiale che istiga un collega a torturare qualcuno debba essere punito con una pena minima di sei mesi e una massima di tre.

già evidenziato un elemento di dubbio molto forte che in quel caso ci fece comunque esprimere un voto favorevole sul provvedimento, ma rimase da parte nostra dubbio di introdurre questo reato nell'ordinamento italiano, non immaginandolo come reato proprio, ma come reato comune e, quindi, in qualche modo modo contravvenendo alla Convenzione dell'ONU del 1984 e anche a quanto accade in molti ordinamenti di altri Paesi. Ebbene, già quello era un punto di grande perplessità ed è evidente che dal nostro punto di vista

Noi pensiamo che sarebbe stata molto più corretta la dizione in cui si faceva riferimento alle «sofferenze fisiche o psichiche», appunto quelle richiamate dal testo della Convenzione dell'ONU; dell'ONU; parlare oggi di «reiterate violenze» e «verificabile trauma psichico» ci sembra un modo per rendere meno individuabile la fattispecie della tortura ed è il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento

rispetto all'accertamento delle condizioni nelle quali avvengono questi atti che definiamo tortura.

se leggiamo il testo, c'è una differenza abissale rispetto a quello che ha letto il Sottosegretario. La normativa internazionale dice cosa è la tortura: quando si prende una persona e la si sottopone - come è nell'immaginario collettivo e nei film - a tutta una serie di violenze per farle confessare qualcosa per farle dire qualcosa, e ognuno immagina tutte le tecniche che vengono utilizzate. Cosa è, invece, la tortura secondo questo testo? Lo rileggo per avere la consapevolezza di quello che votiamo.

e il reato scatta anche se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso. Quindi introduciamo una norma che riguarda minacce

tra questa accezione di tortura e la tortura che vogliamo introdurre nel nostro ordinamento, che tutti abbiamo in mente, ossia una cosa gravissima, che una persona sottoposta a custodia, o sequestrata da un privato o in mano alle Forze dell'ordine o alla magistratura, subisca determinati comportamenti. Torniamo all'ambito psichico. Per voi la minaccia può determinare pressioni psichiche che - il relatore ci dice - devono essere poi esaminate dalla scienza medica per capire se effettivamente il turbamento psichico che viene denunciato è vero o non è vero.

è totalmente diversa da quello che la gente si immagina sia la tortura. Non sto parlando di cose teoriche: è sufficiente che prendiate il testo e lo leggiate per come è stato scritto per rendervi conto che ciò che introduciamo nell'ordinamento è una cosa mirata a

Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti che questo provvedimento è stato approvato da quest'Assemblea a larga maggioranza; è stato poi modificato alla Camera e la Commissione giustizia ha ricostituito il testo votato dal Senato. Mi chiedo se non sia il caso di lasciare solo l'emendamento dei relatori 1.254, che si muove nella stessa linea votata in Commissione, e di ritirare tutti gli altri emendamenti. Infatti, se abbiamo scelto una linea, votata a larga maggioranza da quest'Assemblea, credo che oggi non potremmo smentirci votando emendamenti che aggiungono o modificano piccole espressioni. Il testo, così com'è, fa anche luce su quelle che sono state dichiarazioni in sede di discussione generale, perché ricostruisce, come ha ricordato il relatore, il presidente D'Ascola, quella che è stata la scelta della Commissione e di quest'Assemblea: reato comune con l'aggravante per i pubblici ufficiali. Credo che questa sia la scelta più saggia, se volete farla, altrimenti andiamo a votare, dopo di che vedremo, perché ovviamente se fosse modificato il testo votato dal Senato, probabilmente non ci sarebbe la stessa maggioranza che si è prodotta in prima lettura

Signor Presidente, in linea con le considerazioni espresse dal presidente relatore D'Ascola, vorrei brevissimamente dire che i pareri sono finalizzati al raggiungimento di maggiori coerenze sistemiche, ad evitare

dei pareri espressi dal relatore. È evidentemente nei suoi poteri e ne prendiamo atto. Però vorrei dire una cosa molto chiara a tutti i senatori di questa Assemblea. Questo provvedimento, similarmente ad altri,

Così è accaduto nella stesura del primo testo approvato dal Senato e questo si è verificato anche per la stesura del testo che ha modificato quello della Camera e che viene oggi presentato al Senato. L'azione di Forza Italia, che non è mai stata ostruzionistica in Commissione giustizia né in Aula, si è fatta valere in diversi e molteplici provvedimenti che qui in Assemblea sono passati a larghissima maggioranza. Vorrei essere chiaro su questo punto.

politico: se gli accordi raggiunti in Commissione vengono poi stravolti in Aula, noi non possiamo che prenderne atto e evidentemente, signori senatori, trarne le dovute conseguenze sul piano politico.

il Gruppo di Forza Italia non stipulerà più alcun accordo con la maggioranza in sede di Commissione, con tutto quello che ne consegue con riferimento a molteplici e diversi provvedimenti. In Commissione questo provvedimento è stato varato quasi all'unanimità, ma si è votato un testo che prevedeva la pena minima di tre anni, che adesso si vuole portare a quattro, e che prevedeva anche la parola «reiterate» che invece adesso, sulla base di un emendamento, si vuole oggettivamente eliminare.

così evidentemente confondendo - non so con qual conoscenza del diritto - il reato di tortura con altri reati che andavano contro l'incolumità personale.

bisognava fortificare il concetto che non erano sufficienti un'unica violenza e un'unica minaccia per realizzare e concretizzare il reato di tortura. Dopodiché, questo è quanto volevamo dire con molta franchezza all'Assemblea:

bisogna chiarire i termini della questione. D'altronde, qualsiasi senatore può farlo sol che legga il testo del delitto di tortura nella colonna di sinistra Il termine «reiterate» non è mai esistito in quella fase; ossia, la Commissione giustizia, presieduta dal senatore Palma, ha licenziato, con l'accordo della componente Forza Italia, il testo del delitto di tortura senza inserire il termine «reiterate», come ognuno può

contenutistici e seri, non soltanto per reclamizzazione dei fatti - e abbiamo ritenuto che il termine «reiterate» prefigurasse il rischio di una sorta di delitto abituale, e cioè che dovesse avvenire reiteratamente nel tempo, il plurale «violenze» o «minacce» fosse sufficiente ad affermare quello che io avevo già detto, cioè la necessità che vi fossero più condotte di violenza o di minaccia. Ebbene, per la eliminazione del «reiterate»,

Quest'affermazione è enfatica e, tutto sommato, poteva non esserci, perché è chiaro che chi tortura opera al di fuori dei poteri e doveri che gli vengono attribuiti. Ci mancherebbe altro che si possa ipotizzare una norma di diritto pubblico che stabilisce che un pubblico ufficiale può torturare qualcuno. Ciò nonostante, ci siamo posti il problema - ecco il dare conto all'Assemblea e lo spiegare le riflessioni che vi possano essere delle sofferenze inevitabilmente connesse all'esecuzione di attività coercitive tipiche del pubblico ufficiale e che si possano porre dei casi si lamenta di essere stato torturato per l'esercizio di un potere pubblico e per l'adempimento di un dovere connesso alla sfera pubblica.

Se qualcuno vuole un momento di notorietà provocando, lo faccia pure, ma per me è completamente indifferente. Nella logica che stiamo adesso iniziando a rappresentare, più mi interrompete più perdiamo tempo. Sotto il profilo parlamentare, quando un Gruppo politico si irrigidisce, i senatori del Gruppo di maggioranza, o pseudo-maggioranza, devono semplicemente stare zitti e avere la pazienza di ascoltare. Signor

il quale ha detto delle cose anche condivisibili sul piano giuridico. Ma io non avevo posto un problema di merito in ordine agli emendamenti. Io avevo posto un problema politico

e perché in Commissione non sono stati posti questi problemi, in considerazione della serena collaborazione che si stava sviluppando? Questo è il problema. Poi, se i termini «con violazione di doveri», «reiterate» e via dicendo siano termini migliorativi o peggiorativi a me importa poco, perché abbiamo avuto tutto il tempo in Commissione per affrontare queste problematiche. Ci sembra addirittura singolare che, dopo l'accordo in Commissione, si modifichi il tutto. L'emendamento 1.200 è soppressivo. Noi avevamo immaginato di poter ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 1, proprio in uno spirito di serena collaborazione;

ho spiegato bene perché il termine «reiterate» è stato inserito nel nuovo testo, proprio alla luce della modifica e del ragionamento ideologico che era il presupposto della modifica avvenuta alla Camera. Per noi il termine «reiterate» è assolutamente fondamentale, come è assolutamente fondamentale la pena, che deve essere delimitata in un recinto generale di ragionevolezza, con riferimento al sistema sanzionatorio del nostro codice. Davvero non riesco a comprendere la ragione per cui si ritiene così importante passare da un minimo di tre anni ad un minimo di quattro anni, quando nella realtà sappiamo tutti che la cosa che conta è il massimo di dieci anni. Dobbiamo passare ad un minimo di quattro anni perché, attraverso il giudizio abbreviato e l'eventuale concessione delle generiche, comunque dobbiamo schierarci su un tetto di pena superiore ai due anni e così essere certi di assicurare il carcere a chi commette tale tipo di reato? Ma, signori miei, la dovete finire di aumentare i minimi delle pene e così di dimostrare in modo palese la vostra sfiducia nei confronti dell'agire dei magistrati. Alzare i minimi delle pene significa esclusivamente questo: cari magistrati, voi, quando quantificate la pena che in concreto andate ad irrogare, quantificate sempre la pena in modo troppo basso e costringete noi legislatori ad intervenire per aumentarla, perché non abbiamo più fiducia in voi. Ma dimenticate una cosa, assolutamente fondamentale nel sistema sanzionatorio: i minimi delle pene non particolarmente alti

per irrogare in concreto una pena ragionevole nei confronti di un reato sì odioso, ma che può essere minimale rispetto alle altre tipologie di reato e alle altre tipologie di fatto che possono concretizzare lo stesso reato.

Ve l'abbiamo spiegato qui in

avviene per l'omicidio stradale, ed ora avviene anche per la tortura. Ci sono torture che meritano non dieci anni, ma probabilmente molto di più; ma ci sono dei reati di tortura che devono essere puniti in quanto tortura, ma che richiedono un atteggiamento sanzionatorio di tipo diverso. Alla luce di Alla luce di come si sta prospettando il testo, voi comprendete bene che noi non siamo disponibili a favorire il a favorire il varo di un testo che presenta, dal nostro punto di vista, delle anomalie sia sul piano sanzionatorio sia sul piano della ricostruzione del fatto da parte dell'autorità giudiziaria. È chiaro che quando si scrive «con violenze o minacce» si fa riferimento quanto meno a due comportamenti, e cioè non si fa riferimento a uno schiaffo ma quanto meno a due schiaffi. Ma quando abbiamo inserito «reiterate» abbiamo immaginato un qualcosa che non avesse una sua dimensione temporale minima, ma che avesse una dimensione temporale estesa nel tempo, perché solo se estese nel tempo le minacce e le violenze possono portare a quel turbamento psichico a cui prima si faceva riferimento, così come possono portare alla realizzazione del reato di tortura.

non c'è neanche bisogno della querela di parte.

che, collegata alla minaccia, diventa una spada di Damocle irresponsabile di cui non c'è traccia nelle convenzioni internazionali. Ma dove è scritto, nelle convenzioni internazionali, che un pubblico ufficiale può finire sotto processo per tortura per una minaccia grave

Per me era insoddisfacente, ma per Forza Italia era soddisfacente in quanto riteneva che il testo arrivato in Assemblea, fra spinte e controspinte e rispetto alle cose incredibili scritte alla Camera, fosse comunque un compromesso accettabile.

anche gli atteggiamenti colposi, e non soltanto quelli dolosi. E continuano a ripeterlo in quest'Assemblea, criminalizzando in anticipo ogni azione di polizia o dei carabinieri condotta in difesa dei cittadini. Ciò induce carabinieri e poliziotti ad adottare grande prudenza quando devono intervenire.

Anche quando essi vengono assolti, infatti, vengono criminalizzati da una certa area che ritiene poliziotti e carabinieri, per principio, dei nemici da abbattere. Con questa norma, e non votando questo emendamento, noi apriamo la strada

di realizzare accordi per avere un prodotto legislativo che possa essere condiviso da larghe maggioranze. Proprio in questa ottica, vorrei ricordare che quando il Gruppo di Forza Italia volle soltanto proporre una piccola modifica al primo provvedimento svuota carceri, il Presidente della Commissione giustizia, che pure apparteneva a Forza Italia, votò contro l'indicazione del partito, proprio perché bisogna mantenere l'equilibrio tra quanto si fa in Commissione e quanto si fa in

Eppure avevo chiesto di non ritirare l'unico emendamento dei relatori che si muoveva nella logica introdotta in Commissione. Ebbene, anche quello è stato modificato con il parere del relatore.

Allora mi domando qual è la logica? Che cosa è successo? C'è la volontà di aggregare qualcuno in maggioranza per cui si è cambiata questa logica di voto?

generale, eventualmente sospendendo per un attimo i lavori dell'Assemblea, perché ci sia la possibilità di trovare la soluzione e non perché sia necessario avere il nostro voto.

e convinzione sui cittadini se hanno un forte sostegno parlamentare. Forse a voi non interessa e vi basta un voto di maggioranza. Questo è sbagliato.

quelli che vogliono togliere la parola «reiterate». Sorprende anche noi, perché non si comprende quale possa essere stato il percorso che oggi ha portato a una diversa valutazione su questi emendamenti.

Il "reiterato" è insito, perché la condotta che integra un'ipotesi di tortura, anche pensandolo nel diritto naturale, in un'ipotesi

questa modifica, che non solo incide sugli elementi costitutivi del reato, ma anche sulla pena. Della pena stessa abbiamo discusso; lo si vede anche semplicemente confrontando i testi, quello uscito dal Senato in prima lettura, quello della Camera e quello attuale, emerge che è stato volontariamente deciso di prevedere una pena della reclusione da tre a dieci anni. Non si comprende la giustificazione per la quale adesso debba essere innalzato il limite della pena.

di sospendere l'esame di questo provvedimento, per cercare di trovare delle soluzioni che vedano, su un reato così delicato, la massima unità del Parlamento. In proposito, presidente

Senatore D'Ascola, l'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 191 del codice di procedura penale, inserendo il comma 2-*bis*, che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante tortura; ma non vi è una previsione di alcuna regola o di alcuna norma di coordinamento tra lo svolgimento del procedimento nel quale sono rese le dichiarazioni o assunte le informazioni e lo svolgimento

determinate dichiarazioni ai fini dell'accertamento dei fatti e dell'affermazione della responsabilità, queste dichiarazioni possono essere utilizzate soltanto se non si configura l'ipotesi del reato di tortura, nel senso che non sono state rese sotto tortura. Per arrivare a questo a questo dato, si rende necessario sospendere il processo nel quale le dichiarazioni devono essere utilizzate per attendere l'esito del processo sulla tortura. Lei, presidente D'Ascola, e noi riusciamo ad immaginare quante denunce di ipotesi di dichiarazioni estorte sotto tortura saranno fatte saranno fatte al solo scopo di vedere sospeso il procedimento in cui le dichiarazioni devono essere utilizzate?

tutto, è correggere ulteriormente questo aspetto che vi ho segnalato, che non mi sembra roba da poco. Parliamo di una questione estremamente importante: con le denunce di tortura, potremmo vedere paralizzati tutti i processi nei quali queste dichiarazioni devono essere utilizzate. Ma la richiesta ha anche una finalità politica e in ciò mi riallaccio a quanto dicevano il senatore Palma e la senatrice Stefani.

una convergenza, dall'altro potrebbero realizzare una divergenza. Per queste ragioni insisto affinché i relatori chiedano la sospensione dell'esame di questo provvedimento.

Signor Presidente, il suo ultimo intervento mi agevola in quello che vorrei dire. Abbiamo ascoltato anche il senatore Falanga, che

sia rinviare il dibattito su questo argomento alla prossima seduta, quindi immagino alla prossima settimana, perché, come lei ha già detto, i tempi non sono compatibili neanche con le richieste di intervento su questo singolo emendamento.

non ci si renda conto che, dopo un lavoro fatto in Commissione (a quanto ho ascoltato dai senatori Caliendo e Palma), con tanta leggerezza, quasi da dilettanti allo sbaraglio,

poi si accettano emendamenti che avrebbero sconvolto un accordo più o meno generale già assunto! Politicamente è un atto grave ed è assurdo che si ripeta ciclicamente, perché quando si intende far prevalere

il quale ha illustrato, dal suo punto di vista, la necessità di prenderci del tempo per rivedere ed eventualmente emendare il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, quello relativo alle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante la tortura. Occorre forse ricordare ai colleghi, all'Assemblea e alla Presidenza che l'articolo 2 non è stato oggetto di modifiche alla Camera, ha già avuto la doppia approvazione e quindi, anche volendo, non potremmo più intervenire in sede emendativa. Nel merito, sulla richiesta formulata di

di tirare giacche, fare occhiolini o, diversamente, di voler quasi intimidire gli appartenenti alle Forze dell'ordine, la cui vicinanza da parte del Movimento 5 Stelle è sempre stata oggetto di azioni politiche di difesa, ad iniziare dalle loro condizioni di lavoro e dalle strumentazioni di cui sono dotati.

Il senatore Palma era il presidente della Commissione giustizia e chiude degli accordi a nome di Gruppi parlamentari in Commissione.

ma sono soddisfatto di come questo Governo non incontri più il favore degli italiani. Ora, se vi comportate in questo modo, se fate gli accordi in Commissione

Noi siamo all'opposizione senza se e senza ma e aspettiamo il *referendum* di ottobre sperando che almeno su una cosa Renzi mantenga la parola. Prima ha personalizzato il *referendum* e poi ha detto che smetterà di fare politica. Quando vincerà il no al *referendum* di ottobre, tutti noi aspetteremo gli atti conseguenti e metteremo fine a un atteggiamento nei confronti del Parlamento che non è più accettabile.

Altro che l'obiettivo dichiarato, che non verrà raggiunto, di passare al monocameralismo! Alla fine perderete anche quei pezzi di Governo,

Francamente questo modo di procedere impedisce a noi dell'opposizione di dare un contributo per migliorare alcuni provvedimenti che potevano nascere sotto un auspicio assolutamente diverso.

Presidente, noto anzitutto che, sulla legittima richiesta del rappresentante del Movimento 5 Stelle di procedere alla votazione elettronica, vi è stato l'appoggio. Tuttavia, siccome è marmorizzato nel tabellone, mi chiedo se quell'appoggio sia ancora attuale

del senatore Marin, ma principalmente - senza nulla togliere al senatore Marin - del senatore Caliendo, sono costretto a chiederle la votazione per parti separate

Se non ho male interpretato il pensiero dell'onorevole Caliendo, ho la sensazione che, al di là delle ragioni politiche ampiamente espresse in precedenza,

Presidente, esiste un sito che propaganda il voto per il sì. Ovviamente riporta nomi di illustri personaggi che sostengono il sì al *referendum* costituzionale del prossimo autunno: Giorgio Napolitano, la presidente Finocchiaro e il nostro collega, che non si è mai visto in questa sede, Renzo Piano,

Presidente, è evidente a questo punto che chi gli ha dato il suo appoggio deve temere di essere a sua volta rimosso, e mi auguro solamente dal *web* e non dal globo terracqueo. Ciò, però, dà l'idea della serietà con cui questa persona sta affrontando il *referendum* del mese di ottobre. Utilizza a suo uso e consumo l'immagine delle persone, pensando che i cittadini abbiano l'anello al naso e vadano a votare semplicemente guardando il più bello, come fosse una *soap opera*. Da ultimo, signor Presidente, la prego di tenere conto e di sollecitare la definizione dei tempi e dei modi con cui i comitati possono accedere al servizio radiotelevisivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi abbiamo avuto un confronto sull'informativa del ministro Gentiloni Silveri sulla strage di Dacca, a cui ha fatto seguito un dibattito che ha incluso il gravissimo episodio avvenuto a Fermo, con l'uccisione di un giovane africano per mano di un assassino di casa nostra con evidenti moventi razzisti. Ritengo che non tutti gli interventi siano andati nel senso della responsabilità istituzionale, che per me assume oggi un ruolo fondamentale a tutti i livelli: da quello parlamentare fino al livello territoriale. Anche un consigliere comunale è un pubblico ufficiale e rappresenta la collettività. Ora capirete il perché della mia focalizzazione sul locale, attraverso la lettura di una pubblicazione su un profilo Facebook, che recita: «Questa è una delle vittime italiane a Dacca. Mesi fa, dopo l'attentato di Parigi, pubblicava orgogliosa la sua firma alla petizione su Change.org. Il destino a volte è beffardo e ha voluto che finisse trucidata da dei "bastardi" perché non sapeva i versetti del Corano». Così il neoconsigliere di maggioranza del Comune di Novara Ivan De Grandis, di Fratelli d'Italia, commenta sui *social* la morte di un'italiana per mano dei terroristi dell'ISIS a Dacca. Adele Puglisi, dopo gli attentati di Parigi, aveva sostenuto dal suo profilo Facebook la petizione contro il direttore di «Libero» per la nota prima pagina del quotidiano dal titolo «Bastardi Islamici». Si parla di linguaggio d'odio e di incitamento all'odio razziale, un tema che riguarda da vicino non solo i giornalisti, ma l'intera *agorà* reale e virtuale che investe tutti noi; un tema su cui anche gli insegnanti, che spesso vengono invocati nell'attivare processi educativi - lo abbiamo fatto anche stamattina - sono soli e non possono affrontare da soli la battaglia, se non è comune. La vicenda ieri è arrivata alle cronache nazionali, suscitando sdegno e proteste. Da parlamentare novarese, anche in qualità di componente della Commissione diritti umani, ho stigmatizzato, tra l'altro senza neppure citare l'autore, questo modo di fare politica privo della minima responsabilità, del dovuto rispetto, ma anche di un minimo di empatia, oltre che di buongusto. Avevo invitato il sindaco neoeletto, esponente della Lega Nord, a prendere le distanze da quelle dichiarazioni; un appello rivolto da più parti, soprattutto da tantissimi novaresi che non si riconoscono in quelle parole scritte da un rappresentate istituzionale della comunità. Ebbene, né il sindaco né tantomeno la giunta hanno affrontato l'argomento; neppure un minuto di silenzio per le nove vittime di Dacca, chiesto e ottenuto da una consigliera democratica ieri sera al primo consiglio comunale. Il primo cittadino si è limitato a qualche commento sui giornali locali di questa mattina dove invitava De Grandis a chiedere scusa «se ha urtato» - solo le sue parole - «senza volerlo la sensibilità di qualcuno». Non male per chi si è presentato ai cittadini come «il sindaco di tutti». Peggio, molto peggio di lui il deputato novarese Gaetano Nastri, guarda caso dello stesso partito del consigliere De Grandis. Nastri, da autentico onorevole, ha dichiarato che «le polemiche strumentali mancano di rispetto alla vittima più ancora del *post* contestato»: un insulto senza mezzi termini a tutti, senza distinzioni, coloro che si sono permessi di eccepire. Quello che succede nelle ultime ore a Novara, onorevoli colleghe e colleghi, è sintomatico di quanto i nodi del populismo becero giungano presto al pettine. Giocare sulla protesta per per emergere in campagna elettorale può certamente premiare, ma i risultati sono questi: creare un solco profondo tra il sentire comune e le istituzioni. Parliamo di valori, di identità, di umanità.

Caldara. La città di Novara aveva organizzato una marcia di solidarietà assieme alla comunità islamica per dire no al terrorismo. Novara è la città che si è stretta attorno alla famiglia della dottoressa Rita Fossaceca, impegnata sul fronte umanitario in Kenya dalla parte dei bambini e barbaramente uccisa mentre difendeva la madre da un commando

come questi non siano banalizzati nemmeno quando si usa il *web*. Certi messaggi non possono passare. E, dopo l'intervento di stamattina del Capogruppo della Lega, acquista ancora più valore ricordare la scelta di Adele Puglisi, che si è opposta da cittadina libera al linguaggio d'odio che semina intolleranza, intolleranza, preludio spesso di violenze inaudite. Per questo, proprio stamattina è importante che emerga forte e chiaro da questi banchi la piena solidarietà agli altri otto italiani di Dacca, ma anche a Emmanuel, morto in Italia per mano dello stesso odio che ci fa scrivere sui giornali «Bastardi Islamici». ho già fatto alcuni interventi sul tema dell'acqua

partecipazione popolare. I fiumi sono la culla della civiltà, sono assolutamente indispensabili per la nostra sopravvivenza, sono una delle poche fonti di acqua dolce e, quindi, vanno trattati nella maniera migliore possibile. Esiste uno strumento, che si chiama contratto di fiume, che è un esempio di democrazia diretta dal basso; ha già trent'anni di vita come strumento normativo

C'è un progetto che si sta portando avanti, il contratto di fiume Meolo Vallio Musestre, che è talmente buono che gli è stato dedicato un bellissimo *reportage* televisivo in prima serata su Raitre, all'interno della trasmissione «Scala Mercalli». di un progetto sul quale molti cittadini si sono spesi, attivisti e non, di qualsiasi colore politico, perché è assolutamente eterogeneo, ma che si è interrotto verso la fine dell'anno scorso per motivi ad oggi sconosciuti.

5 Stelle li hanno interpellati in questi mesi, ma non hanno ricevuto alcuna risposta sul perché, la procedura per implementare questo contratto è bloccata. Quindi, ufficialmente il motivo è sconosciuto,

A qualcuno non piace che i cittadini possano avere maggiori poteri di indirizzo nella gestione di un bene così importante come il fiume. E per non far nomi, dico chiaramente che questo qualcuno potrebbero essere i consorzi di bonifica. Qualcuno teme forse per qualche piccolo o grande potere personale? Si preoccupi e continui a temere perché noi, come Movimento 5 Stelle, continueremo a chiedere l'implementazione di questo progetto di democrazia partecipativa dal basso

non sono riusciti ad arrivare, perché il loro mezzo è rimasto in avaria.

Sicuramente quei mezzi dovevano essere rinnovati e sicuramente l'amministrazione è al corrente dei fatti. I mezzi dei vigili del fuoco vanno riparati e, se troppo vecchi, vanno sostituiti. Attendiamo anche noi, e concludo, insieme alle rappresentanze dei vigili del fuoco, una risposta seria e responsabile, perché non è accettabile che quanto è successo debba succedere ancora.

Guarda caso, proprio quando abbiamo un'azienda statale che funziona, cosa fa questo Governo che, come abbiamo sempre detto, è delle banche, il Governo che, anziché fare provvedimenti per aiutare i cittadini contro Equitalia, per aiutare i cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese,

sa per quale motivo. A questo punto a me viene in mente una cosa: forse perché stava dando fastidio al mercato finanziario? Forse perché stava dando fastidio a chi finanzia il Partito Democratico indirettamente attraverso le fondazioni bancarie di Renzi? Presidente, qui ci troviamo allora in uno Stato dove non comanda più il cittadino, ma le banche. Non è possibile avere un Partito Democratico che viene telecomandato dalle banche e - aggiungo - dalle assicurazioni. *(Applausi della

Vorrei parlare di un uomo, Emmanuel Chidi Namdi, per sottolineare che è stato ucciso per razzismo. Oggi l'Italia è in lutto. Tra l'altro, fuori da qui, sui giornali, si parla moltissimo fortunatamente di questo fattaccio, un omicidio che non è solo un atto di violenza contro un essere umano che ha la pelle di un altro colore e vive in un altro Paese. È un omicidio contro i valori su cui si fonda il nostro Paese. È un omicidio contro la storia e contro il futuro. Il futuro - come chi racconta le grandi tendenze dello sviluppo del Pianeta - sarà sempre più fatto di mobilità di persone, che si sposteranno da un Paese all'altro, da un continente all'altro. Erigendo muri, anche ideologici, non faremo altro che rinchiuderci in una prigione dentro la quale diventerà impossibile vivere. Oggi uomini e donne si trovano davanti a una grande sfida, che è una sfida politica: costruire un Paese capace di stare bene dentro il presente e il futuro; un presente di mobilità delle persone e un futuro che sarà sempre più di incontro di diversità; un futuro in cui non deve venire mai meno il rispetto per i diritti umani. I colleghi della Lega - ho sentito stamattina il senatore Centinaio - sono persone responsabili. Per questo mi rivolgo a loro per dire che certe tesi, di fatto, alimentano l'odio e il risentimento verso l'altro, verso il diverso e lo straniero. Alla fine tali ragionamenti generano il terreno di coltura in cui maturano gesti come quello che ha portato alla morte di Emmanuel. Il collega Centinaio poc'anzi ho operato una generalizzazione, mischiando nella categoria "assassinio" aggressioni e omicidi di tipo diverso e facendo esempi per la pena, con questo omicidio che è stato perpetrato per razzismo. È razzismo la peculiarità dell'omicidio del signor Chidi. E non è la prima aggressione razzista in Italia: alimentare l'idea di un'invasione dei nostri Paesi, consentite dal lassismo dei Governi, genera non solo un consenso avvelenato dal risentimento, ma anche l'opinione che le migrazioni piuttosto che gestite possano essere fermate. E questa è un'idea falsa. In definitiva, colleghi della Lega, state ingannando i vostri elettori. State promettendo un futuro che è fuori dalla storia possibile.